apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Informativa

onorevoli senatori, prendo la parola per fare un rapido quanto doveroso punto della situazione sugli eventi che hanno recentemente interessato il personale e le basi della missione UNIFIL in Libano.

poi raggiungerò Bruxelles, dove è in corso un vertice NATO che inizierà stamattina e si concluderà domani. Come ho avuto modo di dire, quella in atto è una crisi gravissima, caratterizzata dal superamento progressivo di diverse linee rosse, nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale. Non da ultima - anzi, per prima - l'Italia, dato che la prima lettera che inviai su questo tema specifico all'ONU, a Lacroix, è datata novembre 2023. Oggi, purtroppo, assistiamo al sistematico ricorso alle armi a Gaza e in Libano, e le vittime sono soprattutto civili inermi già duramente provati dalla pioggia di missili, droni e bombe utilizzati da ambo le parti. L'Italia ha detto e ribadito con chiarezza, non da oggi, che riconosce il diritto di Israele di esistere e difendersi dagli attacchi di chiunque, siano Stati sovrani o organizzazioni terroristiche. Si tratta di un'affermazione e una posizione in cui crediamo e non di prammatica. Allo stesso tempo, con la stessa forza, abbiamo chiesto e chiediamo a Israele di attenersi in modo rigoroso alle regole del diritto internazionale, come della convivenza civile tra Nazioni e Paesi, di proteggere l'incolpevole popolazione civile, a Gaza come in Libano, e di rispettare il personale e le basi, in questo caso di UNIFIL, schierati nel Libano del Sud su preciso mandato delle Nazioni Unite, per l'implementazione della risoluzione ONU n. 1701, che nel 2006 venne varata all'unanimità da tutti i Paesi del Consiglio di sicurezza e sottoscritta sia da Israele che dal Libano. È bene ricordare sempre che Hezbollah, come Hamas, non è uno Stato né un popolo, ma un'organizzazione terroristica, dotata peraltro di una forza militare molto rilevante, che risponde alle logiche militari e politiche di chi non deve rendere conto al proprio popolo. Questa è la realtà dei fatti innegabile. Un ulteriore aggravamento degli eventi, peraltro in parte già in atto, sarebbe però foriero di conseguenze drammatiche per tutti e genererebbe uno scenario che non avrebbe né vincitori né vinti, con incalcolabili conseguenze per il Medio Oriente e probabilmente per gli equilibri mondiali. Per questo motivo, il Governo continua a lavorare per una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, resta l'unica possibile. Lo fa con il viaggio oggi in corso della Presidente del Consiglio in Libano, con le iniziative del Ministro degli affari esteri con una serie di viaggi, chiamate e contatti continui, assidui e quotidiani, che io stesso ho fatto, sto facendo e farò in questi giorni e nelle prossime settimane. Non ultima, proprio ieri, una videoconferenza che ho fortemente voluto con il collega francese con i 16 Paesi dell'Unione europea, che fanno parte dei 50 contributori della missione UNIFIL. Da tale Conferenza è venuto fuori un messaggio unanime e condiviso da tutti: la missione UNIFIL in Libano non solo va rafforzata, ma supportata e, allo stesso tempo, vanno rafforzate e rese credibili le forze armate libanesi, Per dirla in una battuta, servono nuove regole d'ingaggio che puntino a modificare e rafforzare la risoluzione n. 1701, datata 2006, che non solo vanno prese in modo unanime e condiviso, ma devono essere sempre fatte rispettare. A Israele, diciamo con la schiettezza, come si fa tra amici: aiutateci a rafforzare UNIFIL e le forze armate libanesi perché possano svolgere il loro mandato e fare in modo pacifico ciò che avete iniziato a fare adesso con le armi. Veniamo ora ad una rapida descrizione degli eventi più importanti degli ultimi giorni. Il 1° ottobre scorso Israele ha avviato una serie di operazioni militari di terra nel Sud del Libano, con limitate incursioni condotte da unità di ricognizione e sporadici scontri con le linee di difesa della resistenza islamica libanese, in prossimità della *blue line*. Le Israeli Defense Forces (IDF) hanno inoltre sviluppato un'intensa azione di fuoco, colpendo ripetutamente i villaggi di Yarun e Marun Al Ras, nel settore Ovest, e Adassiyeh, nel settore Est, giungendo progressivamente fino alla parte meridionale di Beirut al fine di saggiare l'organizzazione difensiva di Hezbollah, degradare la capacità di comando e controllo e colpire gli *stock* di armamenti di maggior pregio. Per contro, la resistenza islamica ha lanciato centinaia di missili contro il territorio di Israele, per la verità, quasi sempre con effetti trascurabili

dislocate a ridosso della *blue line*, sono arretrate di alcuni chilometri con posizioni in dominio di quota, al fine di non essere coinvolte negli scontri e mantenere una buona conoscenza informativa. Il 6 ottobre scorso, per la prima volta, è stato registrato fuoco di artiglieria e movimenti di unità terrestri dell'IDF a ridosso delle basi avanzate UNIFIL 1-31, 6-50 e 6-52, nel settore Ovest, nonché nei pressi di Blida, nel settore Est. Due giorni dopo, la Marina israeliana ha interdetto l'area al largo del Libano e ha iniziato un'azione di fuoco contro obiettivi ubicati nella fascia costiera. Il 10 ottobre le Forze armate israeliane hanno circondato e osservato con droni la base UNIFIL 1-31, ubicata lungo la *blue line* e occupata da personale italiano. In aggiunta a ciò, le Forze israeliane hanno più volte aperto il fuoco con armi portatili, danneggiando telecamere, sistemi di comunicazione e alcuni serbatoi. Ulteriori azioni di fuoco da parte dell'IDF si sono verificate presso le basi 1-32, presso il quartier generale di Naqoura. Nel primo caso, che ha coinvolto personale italiano, non è stato registrato alcun ferito, in quanto i nostri militari si trovavano già, per ragioni di sicurezza, al riparo nelle postazioni protette nei *bunker*, a seguito dell'innalzamento del livello di *force protection*. Nel secondo caso, è stato invece riportato il ferimento di due caschi blu indonesiani; in ambedue le installazioni era comunque presente anche personale italiano. Sia nel settore Ovest che in quello Est UNIFIL, vi sono stati pesanti scontri tra l'IDF e la resistenza islamica. L'11 ottobre scorso sono state registrate azioni di fuoco dell'IDF contro il quartier generale di UNIFIL di Naqoura, che hanno causato il ferimento di due militari dello Sri Lanka. Inoltre, nella base 1-31 a guida italiana, tre T-wall, componenti modulari del muro di cinta, precedentemente danneggiati, sono stati abbattuti. Nella serata dello stesso giorno il fuoco aereo israeliano, in prossimità della base UNP 5-42, 5-42, occupata da personale ghanese, ha provocato significativi danni infrastrutturali. Il 13 ottobre due carrarmati israeliani hanno fatto irruzione nella base 5-42, con l'intento di recuperare alcuni feriti, sfondando il cancello principale. Dopo un'ora, a seguito delle richieste di UNIFIL, i mezzi hanno lasciato la base. Nel contempo, l'IDF ha condotto molteplici attacchi aerei nella parte meridionale del Libano, colpendo circa 200 obiettivi di Hezbollah. La sera del 15 ottobre, un carro armato israeliano Merkava ha aperto il fuoco contro la base avanzata UNIFIL sotto il comando del contingente spagnolo a Kfar Kela, settore Est, colpendo una torretta della base e danneggiando le telecamere di sorveglianza montate su di essa. Nell'evento non risulta sia rimasto ferito personale delle Nazioni Unite. Al momento, le IDF hanno suddiviso il loro dispositivo militare in quattro settori di responsabilità, a ognuno dei quali è stata assegnata una divisione per un totale di 13 brigate. Sei ulteriori brigate sono attualmente dislocate nella Striscia di Gaza. Tra attacchi e contrattacchi, i due attori principali, Israele e Hezbollah, di cui il legame con l'Iran è evidente e palese, si muovono su un filo sottilissimo e mai come ora il rischio di un conflitto aperto che coinvolgerebbe e forse trascinerebbe l'intero Libano è diventato reale. La scintilla che ha avviato questa nuova fase è stata probabilmente l'uccisione del *leader* politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che stava presenziando alla cerimonia del giuramento del nuovo presidente iraniano Pezeshkian. Ricordo inoltre che gli attacchi israeliani sono stati preceduti da un'inedita operazione condotta attraverso esplosioni coordinate di cercapersone e *walkie talkie*, appartenenti ai membri del Partito di Dio. Ciò ha dato un ulteriore impulso al conflitto, consentendo a Tel Aviv di colpire la *leadership* e ingenerare frustrazione e sfiducia in Hezbollah. Sul piano degli effetti collaterali, i bombardamenti israeliani hanno causato un elevato numero di vittime e feriti tra i civili, che hanno sovraccaricato le strutture sanitarie libanesi e aggravato quella crisi umanitaria che rischia di divenire ancor più ampia di quella di Gaza, che, secondo fonti palestinesi, ha provocato ad oggi oltre 40.000 vittime. Hezbollah, di contro, ha lanciato - ed è una novità - missili balistici a medio raggio verso Tel Aviv, che, seppur largamente intercettati, segnano un ulteriore cambio di passo nelle tecniche di attacco. Negli ultimi giorni sono inoltre emerse alcune vulnerabilità, per la prima volta, nel sistema di difesa aerea israeliano, che hanno presumibilmente indotto gli Stati Uniti all'annuncio di voler schierare una batteria di difesa aerea È chiaro che le azioni israeliane contro le basi delle Nazioni Unite sono state rilevanti e gravissime, come ho avuto modo di dire, violazioni del diritto internazionale e non semplici errori o incidenti. Israele ha dichiarato di aver ripetutamente invitato UNIFIL a lasciare temporaneamente la zona prossima alla *blue line* e di aver chiesto all'ONU di spostarsi più a Nord di circa 5 chilometri per evitare che la missione potesse divenire scudo involontario delle milizie di Hezbollah, che usano le loro posizioni avanzate per proteggersi. Da quanto emerge, tuttavia, dalle dichiarazioni del gabinetto di guerra di Tel Aviv, che mi sono state anche personalmente confermate dal mio omologo Gallant, le azioni israeliane non puntano a occupare la parte Sud del Paese confinante, quanto a ripristinare la sicurezza per consentire il rientro dei circa 80.000 israeliani che sono dovuti sfollare dalle zone di confine con il Libano, implementando, di fatto con la forza, ciò che la risoluzione n. 1701 avrebbe dovuto fare e che purtroppo è rimasta per troppo tempo lettera morta. Subito dopo tali eventi, ho personalmente voluto esprimere al ministro della difesa Gallant e all'ambasciatore israeliano il fortissimo disappunto dell'Italia, richiamando la necessità di astenersi da condotte aggressive contro le forze di UNIFIL. L'ho fatto in modo schietto e accorato, com'è mio costume, consapevole della drammaticità della situazione e del momento che stiamo vivendo. Tali preoccupazioni sono state da me illustrate anche, con uguale forza e convinzione, al vice segretario per le operazioni di pace delle Nazioni Unite Lacroix, che avevo già incontrato e interessato nei mesi passati, rappresentando le difficoltà dell'ONU ad operare efficacemente in un contesto come quello libanese e i rischi conseguenti a queste difficoltà. UNIFIL è una missione complessa, con un mandato di difficile implementazione, regole d'ingaggio inadeguate e forze non equipaggiate per l'attuale situazione del conflitto in essere, ma che, come avevo detto più volte erano già da tempo in questa situazione, quindi non soltanto oggi, che c'è una guerra in quelle zone. Questi presupposti hanno reso l'attuazione di quella risoluzione poco aderente alla situazione sul campo, che è diventata ormai un conflitto tradizionale e aperto. Lo scollamento pratico tra la missione assegnata e la capacità di implementarla rende ora più che mai necessario ripensare e rafforzare UNIFIL, rendendola credibile ed efficace: è l'unica alternativa a una guerra sul campo. Sin dall'inizio della crisi scaturita dagli eventi del 7 ottobre 2023, ho sollecitato una riflessione alle Nazioni Unite per adottare misure concrete e garantire la sicurezza del personale, assicurando nel contempo l'efficacia operativa della missione. Ho voluto anche segnalare la necessità di un incisivo e rapido intervento delle Nazioni Unite che metta UNIFIL nelle condizioni di esercitare una reale deterrenza all'uso della forza. Questo potrebbe essere ottenuto prevedendo diverse opzioni operative, quali ad esempio la presenza di una riserva schierabile rapidamente nel Sud del Libano, garantendo così la piena libertà di manovra delle unità e adeguando l'equipaggiamento in dotazione all'ambiente in cui operano. A prescindere da questo, ad oggi - voglio che sia chiaro e che resti agli atti - non è messa in discussione la nostra partecipazione all'UNIFIL, che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità e fino a quando le Nazioni Unite, insieme ai cinquanta Stati contributori, non decideranno diversamente. Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e minerebbe forse definitivamente la credibilità delle Nazioni Unite. La possibilità della soluzione multilaterale nelle crisi del mondo ha un valore che va al di là del fatto contingente. La presenza dei soldati di UNIFIL può invece ancora costituire un elemento fondamentale per prevenire nuovi e peggiori scontri diretti, nuovi e peggiori conflitti. I caschi blu possono fungere da fattore di pacificazione necessario in questo momento. Inoltre, la loro presenza tornerà ad essere determinante nella fase di stabilizzazione, quando - speriamo tutti molto presto - si potrà abbassare il livello dello scontro. Israele deve comprendere che questi soldati non lavorano per una delle parti, ma sono lì per aiutare a mantenere la pace e promuovere la stabilità regionale. L'imparzialità dei caschi blu è e deve rimanere uno dei pilastri di UNIFIL. Ecco perché le Nazioni Unite non possono accettare di prendere ordini da nessuna delle due parti.

Passando ora alle azioni intraprese dalla Difesa, voglio prima di tutto rimarcare che la priorità mia, del Governo e - presumo - di tutto il Parlamento rimane la sicurezza e la tutela dei nostri militari, del contingente italiano UNIFIL. Sono in costante contatto con il Capo di stato maggiore della difesa, il Comando operativo di vertice interforze e il comandante italiano per monitorare, ora dopo ora, ciò che accade lungo la *blue line*. A giorni, subito dopo il G7 della Difesa, quale, a partire da domani, dedicheremo ampio spazio al Medio Oriente e al Libano, con ulteriori riflessioni e considerazioni, andrò a Beirut e a Tel Aviv. Inoltre, seguirà presto una conferenza in Italia per rendere concreto il sostegno alle forze armate libanesi in termini finanziari, addestrativi e di equipaggiamento. Una prima conferenza virtuale, con la presenza di ben 16 Paesi contributori, si è tenuta ieri, a seguito di un'iniziativa congiunta mia e del collega francese Sébastien Lecornu. Ricordo che oggi la presenza nell'area è molto significativa e che noi contribuiamo con oltre 1.000 militari e con circa 20 unità impegnate a Beirut nella Missione militare bilaterale italiana in Libano, conosciuta come Mibil. Il contingente della Missione bilaterale è stato recentemente ridotto per motivi di sicurezza; ci aspettiamo che possa tornare a operare a pieno regime non appena le condizioni lo permetteranno. Nel frattempo, abbiamo adottato tutte le misure necessarie per gestire i rapidi cambiamenti di situazione, rafforzando le misure di protezione attiva e passiva. Inoltre, i piani di evacuazione sono stati aggiornati e testati e sono pronti ad essere attuati se fosse necessario. Come Difesa siamo pronti a fare la nostra parte e, qualora necessario, in grado di condurre operazioni di estrazione del contingente nazionale e dei nostri connazionali in Libano, anche in modo autonomo. In tal senso, sono già stati preallertati assetti aeronavali per tale scopo e il loro livello di prontezza è stato recentemente innalzato e adeguato alla situazione sul campo. Accennavo prima all'impegno italiano a sostegno alle forze armate libanesi, affinché assumano un ruolo maggiore per la sicurezza e la stabilità del confine israelo-libanese e all'interno del Paese. L'Italia ha sempre cercato di coinvolgere più Nazioni europee, gli Stati Uniti, altre Nazioni e i Paesi arabi in un progetto di assistenza concreta allo sviluppo delle forze armate libanesi. L'impianto iniziale era quello di costituire un fondo internazionale per reclutare, formare, addestrare ed equipaggiare le forze armate libanesi. In questo senso, da mesi stiamo organizzando una conferenza dei donatori necessaria a reperire i fondi per finanziare tali progetti. L'obiettivo è collaborare con i vertici della Difesa libanese per identificare programmi, attività e iniziative mirati a rafforzare le forze armate, permettendo loro di crescere in capacità operativa, credibilità e indipendenza, sottraendole, e sottraendo il Paese, all'influenza di Hezbollah. Con lo stesso spirito, improntato a massimizzare le attività di *capacity building*, stiamo valutando l'ipotesi dell'invio di 200 carabinieri per formare le forze di polizia palestinesi a Gerico. Questa iniziativa risponde a una richiesta avanzata dal segretario di Stato USA Blinken, nella considerazione che gli eventi in Palestina siano estremamente connessi a quanto accade nell'intera area mediorientale. Tuttavia, la sua attuazione è subordinata a una condizione essenziale, che io ho posto: la garanzia totale che tutte le parti coinvolte accettino di buon grado la presenza dei nostri militari. Ritengo che il Libano sia un tassello chiave per la stabilità di tutto il Medio Oriente. Dobbiamo continuare a garantire la nostra piena e costruttiva collaborazione a tutte le iniziative volte a favorire una *de-escalation* della situazione, ma Israele deve comprendere l'importanza di rispettare pienamente il diritto internazionale. In definitiva, l'obiettivo della nostra azione dev'essere quello di stabilire un orizzonte condiviso e delineare un percorso comune per evitare che possa scatenarsi un ulteriore conflitto su una scala sempre più alta in Medio Oriente, con gravissime ripercussioni per tutti. Per questa ragione dobbiamo convincere Israele, un Paese amico, nonostante oggi ne abbiamo censurato alcune condotte, affinché riprenda ad essere un interlocutore con cui dialogare, anche in modo duro, ma con spirito costruttivo, nell'interesse della pace e della stabilità. Non esiste una sola agenda, e non esiste un'agenda che qualcuno possa imporre a tutti gli altri. Le crisi internazionali si risolvono dialogando:

perché accettare che solo la forza e solo la guerra siano il modo di risolvere le controversie internazionali significa negare l'utilità di qualunque organizzazione sovranazionale e multilaterale, e questo noi non lo faremo mai. La mia, la nostra idea, non del Governo, ma vorrei dire del Paese, da cui non recediamo e sulla quale lavoriamo ogni giorno, in modo silenzioso e concreto, è quella di promuovere spazi di pace, rifiutando l'idea che quel territorio sia destinato a un conflitto permanente. L'esperienza ci insegna che, quando una guerra si protrae senza soluzione, poi diventa difficile porvi fine. L'esperienza ci dimostra - io cito sempre l'esempio del Kosovo - quanto sia lungo il tempo con cui poi riusciamo a rimarginare le ferite. Noi siamo in Kosovo da

eppure da venticinque anni siamo in Kosovo e ancora oggi vediamo che quelle ferite non sono rimarginate. Dobbiamo abituarci ad affrontare le crisi internazionali che stiamo vivendo con quest'ottica,

popoli. Dobbiamo partire da questo, che dev'essere non un ostacolo, ma un motivo per partire subito. I tempi e le difficoltà con cui si rimarginano le ferite degli scontri tra i popoli

del Libano, per quanto sia difficile spiegarlo, è necessario che l'ONU non molli e, per quanto sia difficile spiegare la surreale presenza in questo momento di forze militari che non possono agire come dovrebbero, noi sappiamo che una rinuncia sarebbe peggio

dalle due parti. Oggi, da Israele, perché oggi è stato Israele a metterla in difficoltà e, con la schiettezza che si usa con gli amici, gliel'abbiamo detto senza peli sulla lingua: rispettare UNIFIL significa rispettare anche la vostra futura possibilità di avere una pace che non preveda sempre schieramenti di truppe israeliane nel Nord. È un compito che la comunità internazionale ha assunto sulle sue spalle e, certamente, la comunità internazionale deve dimostrare di sapere assolvere.

dall'attuale zona di guerra hanno il diritto di ritornare nelle loro case. È la comunità internazionale che deve garantire la sicurezza degli uni e degli altri nel loro diritto di tornare nelle proprie case. È un compito importante e per il quale occorre unità. Per questo ieri abbiamo messo insieme, in una riunione, 16 Paesi europei e vogliamo farlo nell' ONU. Vogliamo spingere la comunità internazionale ad assumersi sempre di più un ruolo in queste crisi, perché è l'unico modo in cui possiamo affrontare queste soluzioni. L'alternativa sarebbe osservare da fuori scontri sempre più violenti, che non possono che aumentare e coinvolgere altre Nazioni. Parliamo del Libano, una Nazione martoriata dai profughi siriani (sta ospitando più profughi di qualunque altra Nazione al mondo), a cui si aggiungono oggi quelli interni. Se non riusciamo nemmeno in un luogo come quello a trovare la forza di avere un'azione internazionale comune forte, probabilmente non ci riusciremo da nessuna parte. Io non voglio rinunciare all'idea che ci sia la possibilità per il mondo e per le Nazioni, sedendosi intorno a un tavolo, di risolvere in modo pacifico le crisi.

e complessa situazione in Medio Oriente, a cui tutti noi assistiamo preoccupati in questi giorni, mi rendo conto di come la storia tenda a ripetersi e di come, in ultima istanza, le dinamiche umane e le relazioni antropologiche tra gruppi identitari, culturali e religiosi differenti possano condurre ciclicamente a scontri e violenze, con vittime anche civili. Purtroppo questa premessa - permettetemi di dirlo, colleghi - è fondamentale perché, proprio in virtù di questa consapevolezza e dell'attenta analisi del quadro politico, culturale e religioso-identitario di questa bellissima e martoriata terra, occorre calibrare con attenzione, con cautela e in modo ponderato l'azione che l'Italia come sistema Paese intende portare avanti, senza cedere a decisioni avventate proprio sulla scorta dell'emotività. a riprova della grande considerazione di cui godono a livello nazionale e internazionale, portano avanti la loro missione con coraggio, con dignità e con professionalità. C'è un pezzo della nostra Italia migliore lì oggi in Libano, uomini e donne in uniforme che portano orgogliosamente sul braccio il tricolore italiano, ricordando a tutti quello che fa il nostro Paese Paese in quel settore come altrove, ossia contribuire al raggiungimento di una pace giusta, schierandosi con gli alleati e con le organizzazioni internazionali in modo attivo, per far sì che ci sia un cessate il fuoco, che sia assicurato il rispetto del diritto internazionale e che vengano garantite le minime necessarie misure umanitarie. Ben consci delle stringenti regole di ingaggio dettate dalla risoluzione n. 1701 del 2006, che istituì la missione UNIFIL, e consapevoli di quanto la situazione sia divenuta rischiosa, la reazione forse più istintiva e peraltro con buona probabilità ricercata da coloro che hanno perpetrato quegli ingiustificati attacchi su alcune basi dei nostri militari, sarebbe stata quella di ritirare il contingente, e non vi nascondo che il primo pensiero del Governo sia stato e sia proprio quello di garantire la sicurezza ai nostri soldati. In questi casi, però, come in tutte le situazioni più difficili, fermi restando il massimo impegno e la massima accortezza e attenzione nel predisporre i necessari piani di contingenza, monitorando costantemente la situazione e regolando di conseguenza la postura, occorre ragionare e occorre mantenere i nervi saldi, chiedendosi quali siano le conseguenze e gli effetti delle nostre scelte. Ecco che allora rimanere rappresenta il messaggio più potente che al momento si possa dare come Paese, anche se la situazione è difficile, e la missione è per sua natura difficilmente conciliabile con l'ostilità tra le parti. Rimanere significa tenere gli occhi delle Nazioni Unite e quindi del mondo sul conflitto, conflitto, scoraggiare atti di barbarie, limitare, per quanto possibile, reazioni bellicose, proteggere e stabilizzare quell'ormai iconica linea blu che le Nazioni Unite istituirono nel 2006 al confine tra Libano e Israele per conciliare e agevolare una pacificazione tra le parti. Il Governo ha una visione chiara e condivisa sulla complessità dello scenario nella sua interezza, sulla necessità di incoraggiare una soluzione basata sul principio "due popoli, due Stati" quale unico modo per raggiungere un giorno una civile convivenza tra Israele e Palestina, pacificando così l'intera area e disinnescando forme di estremismo e di fondamentalismo. L'Italia c'è e fa la sua parte: da grande Nazione qual è, fa sentire la sua voce con fermezza e risolutezza, in tutte le sue articolazioni, dai suoi coraggiosi soldati fino al Presidente del Consiglio, che si recherà nei prossimi giorni proprio in proprio in Libano per portare quel messaggio di presenza al personale italiano, *in primis*, e a tutti gli altri, dal popolo libanese alle parti in conflitto.

attraverso lei, un messaggio di solidarietà e affetto ai nostri militari impegnati in Libano e in genere in tutto il mondo.

Ci piacerebbe, per esempio, che ci informaste non attraverso i giornali del pensiero di acquistare i sistemi satellitari per le comunicazioni che hanno a che fare con la nostra difesa; non vorremmo leggerlo - appunto - dai giornali, né sapere che sono cose segrete o patti segreti. Bisognerebbe che il Parlamento ne fosse informato

Penso, infatti, che la sua reazione ferma fosse doverosa. Le Nazioni Unite non hanno sempre brillato. Purtroppo, una delle pagine più nere della storia del nostro Continente risale al 1995, al massacro di Srebrenica, che si consumò sotto gli occhi dei caschi blu olandesi. Il rischio che le missioni delle Nazioni Unite risultino inutili o addirittura dannose (perché è chiaro che quando accadono massacri di quel genere sotto i tuoi occhi, ne porti anche tu la responsabilità) è un rischio grave ed è giusto che si lavori per migliorare l'efficienza della missione UNIFIL, perché, signor Ministro, diciamo chiaramente in questi anni è servita a poco; anche le cose che lei ci ha detto oggi sanno un po' dei buoi già scappati dalla stalla. se ci pensiamo, se la risoluzione 1701 del 2006 fosse stata rispettata dal 2006, in questo momento non ci sarebbe probabilmente la guerra tra il Libano e Israele, per come la conosciamo. Se le truppe di Hezbollah fossero rimaste a Nord del fiume Leonte, se non fossero partite decine di migliaia di missili di missili (noi giustamente ricordiamo le azioni di Israele, ma io vorrei sempre ricordare i 12 bambini drusi morti a settembre, vittime di un razzo che arrivava dal Sud del Libano), se se quella zona tra la linea blu e il fiume Leonte non fosse stata occupata da Hezbollah sotto il naso dei caschi blu, probabilmente le cose non starebbero come stanno. il senso del suo intervento, anche quando ha parlato di rafforzare la missione UNIFIL, ha sicuramente una sua logica; davvero rafforzare e in genere poter contribuire al rafforzamento della presenza delle Nazioni Unite e all'importantissima funzione che lei ha giustamente illustrato e e che condivido in pieno, bisogna che alla politica della difesa si affianchi anche una politica estera del medesimo livello: sono due gambe che che devono muoversi in modo sincronico, altrimenti non se ne viene a capo. Le dico la verità: nonostante l'orgoglio per l'azione dei nostri militari, la preoccupazione per la vacuità

perché l'Italia non viene più invitata: è la seconda volta che la presidente del Consiglio Meloni non viene coinvolta in questo vertice con Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti e e questo ci dice di un isolamento e di una difficoltà. Vediamo che il ministro Tajani di fatto è assente, nonostante sia il Presidente del G7 esteri; non c'è uno straccio di proposta italiana, non c'è un ruolo,

l'inefficacia della missione, per come è costruita è sotto gli occhi di tutti, la mancanza di una politica estera incisiva e da protagonisti, ovviamente si tradurrà anche in un maggiore rischio per le nostre truppe. Quindi va bene la missione, se viene ridisegnata; tuttavia, se non saremo autorevoli nello spingere perché venga ridisegnata e rafforzata, il rischio alla fine rafforzata, il rischio alla fine ricadrà anche sui nostri militari.

condivido, e che abbia fatto bene, nel corso dei giorni scorsi, a utilizzare parole molto dure nei confronti di quello che è successo. Ha parlato espressamente di possibili crimini di guerra ha fatto bene, perché l'articolo 8 dello statuto della Corte penale internazionale considera esattamente crimine di guerra l'attacco alle missioni per il mantenimento della pace. Penso quindi che in quel caso abbia utilizzato parole giuste.

qualche giorno fa, e però nel corso dei dodici mesi passati non hanno mai utilizzato questa stessa espressione, crimini di guerra, rispetto a ciò che sta accadendo a Gaza - dove ci sono, glielo ricordo, 42.000 morti nella popolazione civile, 10.000 bambini morti, 7.000 donne morte, eppure da parte del nostro Governo non è mai stata utilizzata in tutti questi mesi, questa definire quelli che Israele sta commettendo a Gaza *(Applausi)* -, poi non ci si può stupire se dinanzi alle parole, in questo caso giuste, che lei ha utilizzato qualche giorno fa, Israele fa semplicemente finta di niente. Termino con una seconda considerazione, che

ore, però, sta accadendo che due Paesi europei importanti e significativi, la Francia e la Spagna, stanno parlando espressamente di sospendere l'esportazione di armi a Israele per evitare che con queste armi Israele continui la sua offensiva e

Dice che è giusto smettere di esportare le armi, come io penso, oppure continua a rifugiarsi dietro questa "faccenda" delle vecchie e delle nuove forniture, che presenta, però, perlomeno dei margini di ambiguità e di poca comprensione? Chiedo

di fatti e di un impegno straordinario per la pace, perché evidentemente la situazione lo richiede fino in fondo.

per il prolungarsi delle ostilità in un'area già martoriata da decenni, per il rischio *escalation* che purtroppo è dietro l'angolo, per la sorte degli ostaggi israeliani, tuttora nelle mani di Hamas dal 7 ottobre, per le vittime civili e per la grave crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. A questo quadro desolante si aggiunge ora la dinamica sul fronte libanese, dove il destino della popolazione civile incrocia rischi e pericoli che pesano sulla missione UNIFIL dell'ONU: una forza di interposizione della quale fanno parte 1.200 militari italiani. Tutti noi conosciamo le ragioni profonde che ispirano la filosofia con la quale le Nazioni Unite hanno articolato il dispositivo di intervento dei caschi blu al confine tra Libano e Israele. Sono le stesse direttrici che giustificano la presenza del nostro Paese quale primo contributore della missione, nello spirito di una Carta costituzionale che ripudia la guerra come risoluzione delle controversie e ci pone, invece, in prima fila per favorire le condizioni della ripresa del negoziato e del confronto diplomatico attraverso la leva del *peacekeeping*. I nostri militari, donne e uomini in divisa ai quali va espressa profonda gratitudine e sostegno, sono messaggeri di pace. Lavorano in funzione stabilizzatrice. La loro presenza si lega alla necessità di mitigare gli impatti umanitari derivanti dalle crisi. Per questo, gli attacchi alle basi UNIFIL avvenuti nei giorni scorsi sono stati condannati con determinazione e hanno trovato compattezza anche nella comunità internazionale. Se questo è il quadro di riferimento, va detto però con altrettanta chiarezza che la missione UNIFIL deve proseguire. Qualsiasi scelta diversa smentirebbe un impegno che si protrae da decenni e non potrebbe che leggersi come l'ennesima debolezza, come segnale di un disimpegno della comunità internazionale dal quadrante mediorientale in un frangente, al contrario, in cui c'è bisogno di maggior protagonismo. Colleghi senatori, io credo che occorra abbandonare certa ipocrisia e chiamare le cose con il loro nome. Al confine tra Israele e Libano si combatte una guerra, ed è giocoforza necessario rivedere le regole di ingaggio della stessa missione UNIFIL; non certo, sia chiaro, per essere parte attiva di un conflitto, ma per consentire ai nostri uomini di agire e di rispondere ai pericoli che si intensificano. In caso contrario si corre il rischio, evidente in queste ore, di essere spettatori in balia degli eventi, privi di qualsivoglia scudo difensivo. Occorre, dunque, sollecitare le Nazioni Unite ad un cambio di registro, per garantire la comunità dei caschi blu e per dotarli degli strumenti attraverso i quali sia davvero possibile adempiere alle funzioni stabilite dalla risoluzione del Palazzo di vetro: in primo luogo, l'attività di disarmo di Hezbollah. Se non si prende atto della necessità di compiere questo passo, si resta nel limbo, nella navigazione in mare aperto nel mezzo di una burrasca. Le vicende di questi giorni chiamano naturalmente in causa questioni più complesse, legate all'evoluzione del paradigma internazionale, ma si riflettono sulle prospettive stesse del sistema incentrato sul ruolo delle Nazioni Unite. Siamo in presenza di una crisi complessiva del modello ONU, evidente dall'incapacità di fronteggiare le sfide dell'oggi e di prevenire quelle future, che pure si stagliano chiaramente all'orizzonte. Le stesse istituzioni multilaterali, a partire dal Consiglio di sicurezza, vivono una crisi profonda, che rispecchia le contraddizioni di questa fase storica turbolenta. Serve un grande innesto di realismo per uscire dalla crisi, abbandonando le ipocrisie, l'ambiguità, ma, scusatemi, anche gli scontri sterili fondati fondati sulle contrapposte ideologie che ci farebbero solo perdere tempo prezioso: in una parola, serve la politica. rappresentanti del Governo, colleghi, ministro Crosetto, innanzitutto desidero ringraziarla, anche da parte del nostro Gruppo, per la sua disponibilità a riferire immediatamente a quest'Aula e tra poco anche alla Camera dei deputati, nonostante la situazione internazionale veda coinvolti i vertici internazionali in riunioni di grande importanza. Approfittiamo della sua disponibilità anche perché giungano al nostro contingente italiano i sensi della nostra gratitudine e preoccupazione per le donne e gli uomini che rendono un grande servizio al Paese, ma non soltanto al nostro Paese. *(Applausi).* Mi permetto un rapido commento alla seconda parte della sua informativa, quella per così dire a braccio, dove ha parlato, metaforizzando, delle ferite che restano dopo un conflitto e che si protraggono per molti anni anche in dipendenza della durata e della profondità

c'è anche il conflitto in Ucraina e mi sembra che lì il nostro atteggiamento sia "fine guerra mai" *(Applausi),* e non la necessità di interrompere il prima possibile quel conflitto. Avremo però altri modi e tempi per parlarne. a ciò che sta accadendo al confine tra Libano e Israele e, più in generale, ciò che sta accadendo da un anno nell'area mediorientale, la prima considerazione che faccio è la seguente. Ci rendiamo conto uno Stato, non un'organizzazione terroristica, che colpisce in modo programmato postazioni di pace, i caschi blu e una missione internazionale? Per quanto ancora Netanyahu potrà abusare della pazienza occidentale? Per quanto ancora noi potremo definirci indignati a parole, ma non essere conseguenti nei fatti? Netanyahu sta portando Israele dalla parte sbagliata della storia e lo sta facendo da un anno. E allora non si tratta soltanto della questione della missione UNIFIL, di quello che sta succedendo in particolare nella base 1-31. Siamo molto preoccupati dai tempi, perché lei ha parlato di una postura diversa della missione, della necessità di incrementare il personale, controbilanciando la retrocessione delle truppe di Israele. Credo che questo sia incompatibile con il tempo e il fatto che il nostro contingente sta usando le razioni K per nutrirsi perché non hanno più approvvigionamenti. Abbiamo una situazione drammatica in questo momento, non nella prospettiva futura. Oggi quello che occorre fare è proporre sanzioni a chi non sta rispettando il diritto internazionale. *(Applausi)*. Noi l'abbiamo fatto nella nostra proposta di risoluzione di martedì in vista del Consiglio europeo. Servono sanzioni economiche, finanziarie, commerciali e diplomatiche nei confronti di un Paese che sta violando il diritto internazionale e che si sta macchiando di crimini di guerra *(Applausi)* per quello che succede oggi sul confine con il Libano e per quello che è successo per un anno nel territorio di Gaza, come ha ricordato molto bene il senatore De Cristofaro. Non è accettabile un'altra postura. Sul tema delle armi concludo, Ministro, dicendo che al di là che l'Istat ha ha reso plateale il fatto che abbiamo continuato a inviare circa 7,6 milioni di euro nei primi sei mesi di quest'anno armi ad Israele, con una valutazione caso per caso, non credo che sposti il tenore del conflitto ciò che stiamo facendo, ma è una questione di postura politica. Noi non possiamo più accettare, non soltanto di consegnare prodotti militari rispetto a contratti precedenti il 7 ottobre dell'anno scorso, noi non dobbiamo più neanche acquistare armi da Israele. *(Applausi)*. Noi dobbiamo smetterla di avere rapporti commerciali con Israele. Esattamente come abbiamo sempre sostenuto la necessità di mettere sanzioni nei confronti della Russia che ha invaso l'Ucraina, io non capisco perché bisogna abbassare la testa e dire che ciò non è possibile con uno Stato che, lo ripeto, si sta mettendo dalla parte sbagliata della storia.

anche nella relazione che ci ha illustrato. In tale momento è di grande soddisfazione notare come il Governo e lei sappiate ben rappresentare il nostro Paese. Ritengo proprio che il Governo italiano abbia dimostrato come, all'interno di un sistema di alleanze occidentali del quale orgogliosamente facciamo parte, sia possibile ribadire anche duramente - e lei lo ha fatto duramente - una ferma condanna ad azioni compiute proprio a danno di un Paese (e voglio utilizzare le parole che lei ha usato) amico ed alleato Le inaccettabili azioni israeliane contro quella missione, la nostra missione internazionale UNIFIL di cui facciamo parte, anche qui orgogliosamente con soldati che portano il Tricolore non solo sul braccio, ma io voglio dire anche nel cuore, non possono in effetti non essere condannate. Anzi, fanno davvero male; fanno male, perché l'Italia con Israele ha sempre mantenuto un rapporto di profonda amicizia, un'amicizia fraterna e di supporto, anche nei momenti più difficili. Io personalmente - tra l'altro assieme ad altri senatori presenti in quest'Aula - mi sono recato in Israele e nel kibbutz di Be'eri, uno dei luoghi dove è avvenuto uno dei più vili massacri compiuti da quei vigliacchi assassini di Hamas, e ho ancora negli occhi i muri butterati dai proiettili, il sangue sulle pareti, le foto degli ostaggi appesi a quello che era rimasto delle abitazioni, ostaggi che purtroppo non sono più tornati a casa. Ho visto anche i video del massacro, che probabilmente abbiamo visto tutti proiettati sugli schermi più volte, e anch'io, come molti altri, ho dovuto distogliere gli occhi da tanta furia di immagini straordinariamente violente. In quel momento, signor Ministro, mi sono sentito appartenere a quell'avamposto occidentale che qualcuno in questo momento vorrebbe cancellare dalla mappa geografica. In quel momento mi sono sentito - devo dirlo con serietà e onestà - israeliano. Proprio per questo la notizia di quell'attacco ai nostri militari mi ha fatto davvero male, proprio perché profondo sostenitore e amico di Israele; come fanno - e qui ribadisco il concetto che lei ha espresso - i veri amici, mi sento di dire le cose come stanno, anche quando emergono errori o gravi incomprensioni. Le nostre truppe sono presenti in Libano meridionale su mandato delle Nazioni Unite, i nostri uomini e le nostre donne operano con professionalità e spirito di servizio e non sono - l'ha detto anche lei, ma lo voglio sottolineare - secondi a nessuno. E la ferma condanna del Governo a queste azioni va proprio nella direzione di cui abbiamo parlato e dimostra come a un'Italia a testa alta nessuno deve permettersi di dire cosa deve fare. Israele è e rimane un Paese amico ed alleato, un bastione di sicurezza in un'area che tutti consideriamo instabile. Con Israele condividiamo valori democratici e strategici, ma proprio perché amico possiamo dire con franchezza quando sbaglia. Condanna all'attacco, sì, lo abbiamo detto con forza, ma è anche importante ribadire, come ricordiamo tra l'altro per altre guerre, che qui c'è un aggredito e un aggressore, e Israele è l'aggredito e Hamas ed Hezbollah sono gli aggressori. Non possiamo far finta di nulla, non possiamo far finta di non vedere la pioggia di razzi che ha colpito Israele dal Sud del Libano. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a chi tiene ancora in ostaggio inermi civili israeliani; e soprattutto non possiamo non collegarli al regime iraniano, altro passaggio importante, quello degli Ayatollah, quello che fustiga le donne e incarcera gli omosessuali, quello stesso regime iraniano e le altre organizzazioni islamiste ad esso collegato, come Hamas ed Hezbollah, che troppi *supporter* hanno nell'Occidente e purtroppo anche in Italia. Questo però ci fa capire forse, una volta di più, come con uno sforzo diplomatico - successivo si spera al vicino cessate il fuoco - si possano appunto rilanciare quegli accordi, i famosi Accordi Abramo, come ha ribadito anche ieri la presidente Meloni, che sarebbero probabilmente il vero fattore di stabilizzazione in questa regione. Una stabilizzazione di questa regione e di questi conflitti avrebbe certamente dei benefici significativi, sia a livello globale, ma anche per la nostra Nazione, con un'auspicabile veloce ripresa di quelle che sono le rotte commerciali navali nel Mar Rosso e il rilancio anche di un altro grande progetto a cui l'Italia tiene moltissimo, che è l'IMEC Indo-Mediterraneo per collegare l'Indo-Pacifico al mar Mediterraneo sul quale, giustamente, il nostro Paese rivendica un ruolo da protagonista. Concludo, Presidente, con una considerazione: lei ha parlato di pace, pace, che ovviamente è auspicabile e - com'è stato detto in quest'Aula - noi lavoriamo per la pace anche attraverso queste missioni. La pace deve essere auspicabile in tutti i teatri di guerra, compreso quello ucraino. sottolineando ancora una volta la nostra vicinanza ai militari impegnati in una missione internazionale probabilmente tra le più complesse,

che ha seguito con il coinvolgimento e nella riunione di ieri, promossa insieme a Sébastien Lecornu, sono il modo con cui si deve procedere nelle azioni internazionali, coinvolgendo tutti i sedici Paesi europei coinvolti nel settore Ovest. L'ho trovato corretto dal punto di vista diplomatico e della capacità di tenere insieme

Ho trovato una caduta di stile il non coinvolgimento del Ministro della difesa spagnolo nella dichiarazione a quattro che ha fatto il ministro degli affari esteri Tajani, anche perché sono gli stessi spagnoli, con il generale Lazaro, a guidare l'operazione UNIFIL, che anche noi abbiamo guidato in questi anni. La stessa presidente Meloni, che bene ha fatto all'inizio con la dichiarazione a tre con il presidente Macron e il premier Sánchez, poi in Aula non ha preso una posizione netta nei confronti del Governo israeliano: non avete inserito nella risoluzione una condanna di quello che ha fatto Israele nei confronti di UNIFIL. Più in generale - lo voglio dire recuperando le parole di equilibrio che abbiamo ascoltato da parte del Ministro della difesa questa mattina - bisogna però essere conseguenti. Spero, ministro Crosetto - glielo dico per il tramite del Presidente del Senato -, che lei queste parole di buonsenso ed equilibrate le possa riprendere in Consiglio dei ministri. *(Applausi)*.

confronti di un Paese amico abbiamo il dovere di non limitarci nelle sedi internazionali, guidando il G7, o quando siamo nelle sedi europee, a dire - come lei pure ha giustamente ha detto - che i caschi blu non prendono ordini da nessuno deve discutere all'interno delle Nazioni Unite): noi oggi abbiamo bisogno di andare oltre, abbiamo bisogno di prese di posizioni simboliche. Per questo non abbiamo condiviso la scelta del Governo di astenersi sulle risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite *(Applausi)* nel momento in cui c'è bisogno di far sentire a Netanyahu che l'Europa è unita. Abbiamo rotto il fronte. Quelli sono i luoghi in cui noi dobbiamo salvaguardare il diritto internazionale e l'importanza del multilateralismo: l'Italia conta se il multilaterale funziona. Oggi l'attacco che mi preoccupa di più è quello di Netanyahu. Hezbollah mi interessa meno perché la condanna è unanime e nessuno mette in discussione che sia un'organizzazione terroristica: c'è una condivisione molto larga in Europa. Non abbiamo a che fare con Hezbollah, evidentemente, ma con Israele sì. È un Paese amico con cui abbiamo accordi di cooperazione e abbiamo il dovere di essere molto netti nel momento in cui c'è un attacco senza precedenti al multilateralismo e al diritto internazionale. Questo è il punto fondamentale che mi aspetto che il Governo italiano, insieme ai Paesi europei, a maggior ragione quando è alla guida del G7, possa portare avanti. Sul punto in sé, sé, penso che dobbiamo fare una riflessione per capire se ci siano le condizioni di sicurezza, in questo caso anche sui duecento carabinieri richiesti a Gerico. Condivido e sottoscrivo le parole del Ministro: si mandano se ci sono le condizioni di sicurezza e le condizioni perché possano operare. operare. Approfitto, nel momento in cui noi chiediamo che vengano garantite le condizioni di sicurezza, per inviare, anche a nome del Gruppo Partito Democratico, la solidarietà e la vicinanza alle donne e agli uomini del contingente UNIFIL. Una riflessione va anche fatta - e a tale proposito dobbiamo dare atto al Ministro, che è stato uno dei primi a sottolinearlo e penso che sia corretto farlo - sulla distanza che c'è tra le finalità del mandato in base alla risoluzione n. 1701, in cui è previsto lo smantellamento di tutti gli insediamenti di Hezbollah nella zona tra il fiume Litani e la linea blu, e le regole di ingaggio che sono state date alla missione UNIFIL per poter mantenere le finalità del mandato. Questo è sotto gli occhi di tutti e penso che l'Italia possa prendere l'iniziativa, insieme agli altri 16 Paesi europei, per adattare le regole d'ingaggio, perché, se li lasciamo lì con le mani legate dietro la schiena e con un mandato con aspettative molto alte, rischiamo veramente di delegittimare una missione che invece è fondamentale e lo è ancor di più per l'Italia, che ha una credibilità enorme nell'area, costruita negli anni dal 1978 in poi. Anche per mantenere quella credibilità quella funzione di ponte verso il mondo arabo, abbiamo l'esigenza di tenere insieme le finalità condivisibili della risoluzione n. 1701 con delle regole di ingaggio che permettano ai nostri di fare il loro lavoro.

tramite lei vorrei rivolgere al ministro della difesa Guido Crosetto un grande apprezzamento per la straordinaria informativa che ha fatto in quest'Aula oggi e che proseguirà alla Camera dei deputati. perché mi richiamo alla conclusione che ho visto nel punto più essenziale e forte, che segna il valore della nostra politica estera e di sicurezza nel mondo. Lei ha detto, signor Ministro, che i nostri uomini in UNIFIL sono lì per una convinzione del Governo Meloni: è l'Italia che fa la differenza con le operazioni di pace in diversi contesti (ONU, NATO, "coalizioni di volonterosi"), nei quali ottiene riconoscimenti così forti da convincere coloro che partecipano ad affidare il comando ai nostri valorosissimi comandanti ed ufficiali, ai quali va il nostro doveroso apprezzamento (ancora oggi bisogna ripeterlo). *(Applausi)*. Sempre tramite il signor Ministro della difesa, vorrei esprimere, da parte del Gruppo Fratelli d'Italia, un'ammirazione per il comandante Stefano Messina e per tutti i suoi uomini e donne impegnati in UNIFIL. *(Applausi)*. Il primo punto che lei ha affrontato, tra i diversi, importanti e spesso sottaciuti punti nei dibattiti parlamentari, parlamentari, è la posizione di assoluta inaccettabilità espressa dal Presidente del Consiglio, da lei e dall'intero Governo per l'attacco subito da UNIFIL; un attacco sicuramente illegale, e che, a nostro giudizio e a giudizio del Governo, viola l'ordinamento internazionale. Ma forse non è stato dato alcun seguito a quelle denunce, a quelle prese di posizione? A posizioni esplicite che anche la risoluzione di maggioranza presentata l'altro ieri in Senato ha incluso nella sua dichiarazione? Non è assolutamente vero, perché il Ministro degli esteri di Israele, proprio recependo queste nostre istanze, le istanze del Governo Meloni, le preoccupazioni e anche la denuncia, mi pare che si sia manifestato in modo chiarissimo. E credo che di questo si debba prendere atto. Il Ministro degli esteri israeliano ha detto: «Israele vede UNIFIL come un'organizzazione che svolge un ruolo importante nel giorno dopo la guerra contro Hezbollah. È l'organizzazione terroristica Hezbollah che usa il personale UNIFIL come scudi umani, sparando deliberatamente ai soldati dell'IDF da posizioni vicine alle posizioni UNIFIL, per creare attriti. Lo Stato di Israele continuerà a fare ogni sforzo per evitare di danneggiare UNIFIL, il tutto coordinandosi con i comandanti di UNIFIL e in conformità con il diritto internazionale». Dal punto di vista personale, signor Ministro, mi permetterei di dare un'apertura di credito, anche da parlamentare, a quello che viene detto dal Governo di Israele, perché sono personale testimone, avendo visitato qualche anno fa i tunnel scavati da Hezbollah al di sotto della linea blu per accerchiare le forze israeliane,

contro militari israeliani, da parte delle autorità e della giustizia israeliane nei confronti di militari che hanno operato a Gaza. L'Italia è in Libano per manifestare la sua fiducia nel futuro delle operazioni di pace e anche nella giustizia internazionale. L'Italia è infatti portatrice di principi di assicurazione alle vittime di una retribuzione certa verso i grandi crimini contro l'umanità e di guerra. Questo è un altro valore d'insieme della nostra presenza in Libano. Su Hezbollah non si parlerà e non si discuterà mai abbastanza nelle sedi politiche competenti, a cominciare - anche se "fuori area" - dal vertice NATO, che è sicuramente un'occasione per

e politicamente equilibrato, non è più sostenibile che due Ministri di Hezbollah all'interno del Governo libanese e una maggioranza guidata da Hezbollah

Le distrazioni, chiamiamole così, i compromessi, li ricordiamo tutti: i Presidenti iraniani venuti a Roma in Campidoglio e ricevuti di fronte a statue romane rivestite da lenzuoli,

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni

Signor Presidente, onorevoli senatori, riguardo alle difficoltà delle imprese italiane produttrici di burro, causate dalle forti oscillazioni delle quotazioni sul mercato europeo, rilevo quanto segue. L'Unione europea svolge un ruolo chiave nel mercato globale del burro, ponendosi come il secondo esportatore mondiale, oltreché uno dei maggiori consumatori. Il mercato del burro risente, nel contesto europeo, delle dinamiche mondiali riferite all'offerta e soprattutto alla domanda. Quest'ultima, infatti, ha registrato un notevole aumento anche a seguito di un progressivo cambiamento delle abitudini alimentari, comportando un significativo incremento delle importazioni, specialmente nei Paesi asiatici. La produzione di burro dell'Unione europea è pari a oltre 2 milioni di tonnellate annue e, dopo la contrazione registrata tra il 2020 e il 2021, è rimasta sostanzialmente stabile nel periodo 2021-2023, registrando tuttavia un'ulteriore riduzione nel periodo gennaio-luglio 2024. Attualmente, a influire sul calo della produzione è la minore disponibilità di latte in alcuni dei principali Paesi produttori, determinata da molteplici fattori quali i cambiamenti climatici, l'aumento dei costi di produzione, le politiche di riduzione delle delle emissioni e, più recentemente, anche le difficoltà legate all'epidemia della lingua blu. Le predette oscillazioni nella produzione stanno determinando tensioni sui prezzi, con i listini del burro in forte aumento nelle principali piazze di scambio europeo. Per quanto invece concerne il contesto nazionale, la produzione di burro si attesta a 93,5 miliardi di tonnellate annue e - a eccezione del calo registrato nel 2022 - è rimasta sostanzialmente stabile nel quinquennio 2019-2023. Il sistema produttivo italiano genera un'offerta di burro che soddisfa poco meno del 63 per cento del fabbisogno interno. La restante quota, provenendo da provenendo da forniture estere, ha reso il mercato nazionale del burro dipendente dalle dinamiche europee e mondiali. Ovviamente, le fluttuazioni dei prezzi nella fase all'ingrosso si sono trasferite in maniera asincrona nelle fasi al dettaglio; in particolare, dopo il picco raggiunto a fine 2022 (12,4 euro al chilo), con oscillazioni in diminuzione tra il 2023 e i primi otto mesi del 2024, si registra una tendenza nelle ultime settimane verso una ripresa dei prezzi che verosimilmente proseguirà. Tale previsione, necessariamente aleatoria, potrebbe sicuramente far supporre interventi speculativi sul mercato che, tuttavia, risultano difficilmente arginabili a livello nazionale. Infatti, occorre tener presente che, come per tutti gli altri prodotti agricoli sottoposti alle regole dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, i singoli Stati membri non possono prevedere misure unilaterali di intervento sui mercati. Qualora la Commissione o altri Stati membri molto più interessati dal mercato del burro, a seguito di produzioni molto più rilevanti di quella italiana, dovessero presentare proposte nel senso prospettato dagli interroganti, l'Italia assicurerà come sempre il massimo impegno a tutela degli interessi dell'intera filiera. Per quanto concerne il contrasto alle pratiche commerciali sleali, ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2021, rappresento che il nostro Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) ha svolto nel 2022 un'incisiva attività di verifica, effettuando sino a oggi più di 700 controlli, molti dei quali nei confronti di operatori del settore lattiero-caseario, ivi compresa la grande distribuzione organizzata. I controlli hanno interessato, in particolare, la verifica delle irregolarità e del rispetto dei contratti di fornitura e le tempistiche di pagamento nonché di condizioni contrattuali di acquisto e di vendita eccessivamente gravose. A seguito di tale attività, sono state oggetto di contestazione per irregolarità numerose infrazioni alla normativa vigente, in particolare in materia di rispetto delle condizioni contrattuali. Tale attività, anche per i prodotti del settore di cui trattasi, sarà rafforzata nell'ambito della programmazione per la prossima campagna di controllo, in considerazione altresì delle nuove previsioni normative introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2024, convertito in legge n. 101 del 12 luglio 2024, con particolare riguardo a quanto stabilito in materia di costi di produzione. Infine, evidenzio che l'istituzione della cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare ha permesso, dall'inizio del 2024, di operare in modo sinergico e coordinato. In tale contesto, le circa 5.000 verifiche effettuate anche nell'ambito del settore lattiero-caseario e sulle pratiche commerciali sleali hanno consentito di rilevare numerose irregolarità e di procedere, nei casi appropriati, al sequestro dei prodotti. Assicuro che il Ministero continuerà a seguire con la massima attenzione la questione per arginare le difficoltà economiche dei produttori di burro, divenuto una risorsa preziosa sui mercati internazionali.

a fronte di molte altre interrogazioni, anche dei nostri colleghi, rispetto alle quali latita ogni tipo di chiarimento da parte del Governo. È chiaro che il tema del burro è solo l'apice di un problema più vasto, che è quello della divergenza tra tra il ricavo percepito dal produttore - cioè dall'allevatore, spesso piccoli allevatori, allevatori di montagna, che producono prodotti di grande qualità - e, il costo che noi troviamo negli scaffali dei supermercati,

da un lato il produttore, l'agricoltore, la famiglia coltivatrice diretta non ricava soddisfazione dal lavoro che fa perché non ha remunerazione e, dall'altro lato, c'è un margine che viene mangiato dalla grande distribuzione, che poi ricade sulle famiglie e sui consumatori. quindi che questo sia un primo banco di prova anche rispetto alla norma introdotta con il cosiddetto decreto-legge agricoltura sulla verifica del costo minimo di produzione, rispetto alla quale noi ci siamo espressi sul principio che si vuol perseguire, cioè quello di determinare un costo minimo di produzione rispetto al quale non si può scendere nell'acquisto del prodotto.

queste oscillazioni di prezzo e intervenire lì dove c'è la speculazione, dove ci sono soggetti che mangiano sul sudore, la fatica e le aspettative di tanti piccoli e medi agricoltori che fanno grande il nostro Paese.

di recente balzato nuovamente agli onori della cronaca, del cittadino americano coinvolto nell'uccisione del maresciallo dei carabinieri Cerciello. Si sottolinea altresì nell'atto di sindacato ispettivo che l'imputato, oltre a beneficiare della consistente riduzione della pena da ventidue a undici anni, applicata dalla corte d'assise d'appello di Roma all'esito del rinnovato giudizio di appello, ha chiesto ed ottenuto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Chiaramente la notizia ha destato sconcerto e, nel contempo, vicinanza alla famiglia della vittima e all'intera Arma dei carabinieri che quotidianamente, come nel caso specifico, affronta elevati rischi per servire il proprio Paese. Si rappresenta che, non appena avuta contezza delle notizie relative ai fatti dedotti dall'interrogante, la competente articolazione del Ministero è stata prontamente incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti. È stata dunque acquisita una dettagliata relazione del Presidente della corte di appello di Roma, che ha ripercorso l'*iter* processuale dell'intera vicenda giudiziaria. Secondo l'aggiornamento trasmesso dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (DOG) il 9 ottobre scorso, la sentenza pronunciata dalla corte di assise di appello risulta essere stata depositata, completa di motivazione, il 23 settembre 2024. Per completezza, è stata acquisita anche l'ordinanza emessa il 25 settembre 2024 dal tribunale per il riesame, confermativa dell'ordinanza cautelare del 15 luglio nei confronti degli imputati, a seguito dell'appello proposto il 16 luglio 2024 dal procuratore generale presso la corte di appello di Roma avverso l'ordinanza del 15 luglio 2024, con la quale la stessa corte di assise di appello di Roma aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti dell'imputato cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo. Analizzando il provvedimento cautelare acquisito, emerge che il tribunale del riesame (cioè il giudice che ha deciso sull'appello avverso il provvedimento che aveva concesso gli arresti domiciliari all'imputato) ha escluso l'applicabilità della doppia presunzione di legge, ovvero della ricorrenza delle esigenze cautelari e della possibilità di soddisfarle unicamente con la misura cautelare di massimo rigore, sulla scorta della seguente testuale motivazione: plurimi elementi sopravvenuti ai fatti, valutati congiuntamente ad altri preesistenti, inducono a ritenere che, nel caso di specie, le esigenze cautelari si siano attenuate e possano dunque essere soddisfatte anche con una misura diversa da quella di massimo rigore. In particolare, il tribunale ha ritenuto di valorizzare elementi specifici quali: la responsabilità penale dell'imputato sensibilmente ridimensionata in quanto da una condanna per concorso in omicidio volontario alla pena di ventidue anni di reclusione, si è passati ad una condanna per concorso anomalo (articolo 116 del codice penale) in tale delitto alla pena di anni nove; il fatto che l'imputato era detenuto in carcere dal luglio 2019 e dunque da circa cinque un periodo di detenzione obiettivamente considerevole; la circostanza che l'imputato non soltanto aveva tenuto in carcere un contegno corretto, ma aveva partecipato attivamente all'opera di rieducazione, risultando dalla relazione comportamentale del 13 febbraio 2024 della casa circondariale di Velletri che lo stesso, oltre ad aver intrapreso in carcere gli studi universitari, si era confrontato proficuamente con gli operatori istituzionali e aveva svolto attività lavorativa, acquisendo sempre maggiore consapevolezza della sua vicenda processuale. Sulla base di tali valutazioni, il tribunale del riesame è giunto alla conclusione che la misura degli arresti domiciliari, tanto più se applicata con gli strumenti di controllo a distanza e con i divieti di comunicazione, comporta una limitazione della libertà di movimento sufficiente a scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie. Peraltro, con riferimento alla diversa esigenza cautelare del pericolo di fuga, è stato sottolineato che la pena residua espianda è prossima alla soglia per l'accesso a misure alternative alla detenzione, per cui, in tale contesto, l'interesse dell'imputato a darsi alla fuga e a sottrarsi alla pena residua risulta notevolmente scemato. va osservato che l'ordinanza del tribunale del riesame, diffusamente motivata, sia in punto di fatto che in punto di diritto, esamina ed affronta tutte le censure sollevate dal pm appellante, anche alla luce dei principi e degli arresti della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. Allo stato, pertanto, non emergono, a carico dei giudicanti della fase cautelare, profili di rilevanza disciplinare per la decisione adottata, attesa l'insindacabilità disciplinare ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 2006, dell'attività di valutazione dei fatti e di interpretazione di norme. Analogamente è a dirsi quanto alle motivazioni della sentenza depositata il 23 settembre 2024 dalla corte di assise di appello di Roma che, dopo aver analiticamente ripercorso lo svolgimento del giudizio ordinario di primo grado, i motivi di impugnazione proposti, i ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di assise di appello e la motivazione della stessa sentenza della Corte di cassazione, ha provveduto in conformità alle statuizioni della suprema Corte sulla valutazione del concorso nel reato di omicidio. Ripercorrendo, inoltre, le censure mosse dai giudici di legittimità alle sentenze di merito, l'organo giurisdizionale di appello ha diffusamente analizzato i principi di diritto che regolano il concorso di persone nel reato e, in tale contesto, l'organo giurisdizionale ha analizzato i principi che regolano quell'istituto e il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo del reato, secondo argomentazioni e valutazioni

nel suo complesso. Stiamo parlando dell'uccisione del maresciallo Cerciello, che nel luglio del 2019 fu ucciso a coltellate da due americani, Lee Elder Finnegan e Gabriel Natale Hjorth, arrestati dopo poche ore. Nel febbraio del 2020 iniziò il processo a Roma, nel maggio del 2021 furono condannati all'ergastolo e al risarcimento di un milione di euro, nel marzo del 2022 la pena fu ridotta

a poche centinaia di metri da qua: una sentenza orripilante, di cui io, come cittadino, mi vergogno e biasimo coloro che hanno preso questa decisione. Avevo chiesto un'ispezione. Lei mi racconta fatti di diritto, ma voglio affermare in questa sede il mio biasimo nei confronti dei magistrati che hanno emesso una sentenza vergognosa,

quest'estate, mentre il maresciallo Cerciello è sottoterra. Queste decisioni offendono gli operatori della sicurezza, l'Arma dei carabinieri, le Forze dell'ordine e le voglio biasimare in questa sede. Altro che ispezione! Andavano cacciati dalla magistratura.

contestato questa sentenza con veemenza adeguata, pari a quella odierna, viene emessa una nota da tale Gaetano Scalise, avvocato, che risulta - così si qualifica, lo sarà - presidente della camera penale di Roma, il quale replica ai miei attacchi. Avrei capito se avesse replicato il magistrato: io sono per la *par condicio* della polemica, se attacco non mi meraviglio che mi si replichi. Ma i magistrati, vili e muti, hanno affidato il compito di rispondere a Scalise. Perché il presidente della camera penale deve rispondere a un parlamentare che attacca dei magistrati? Per avere la benevolenza di quei giudici, quando andrà coi suoi clienti davanti a loro?

Faccia rispondere quelli che stanno, nella vergogna delle sentenze emesse, chiusi nei palazzi. Scalise si vergogni! Perché mi deve rispondere, per quale ragione? Perché deve rispondermi il presidente della camera penale? Si vergognino Scalise e i magistrati. Se fa il fattorino dei magistrati, si dimetta da presidente della camera penale. camera penale. La magistratura ha scritto pagine di vergogna in questi anni. Abbiamo avuto la condanna di De Pasquale, noto persecutore di Berlusconi. Abbiamo avuto la condanna di Davigo, che diceva che esistevano solo colpevoli per i quali non si era dimostrata la responsabilità. Aveva ragione: la frase valeva anche per lui, evidentemente, perché è stato condannato anche in appello. Gli auguriamo assoluzioni in Cassazione. Lei ricorderà che Davigo aveva questa strana teoria: non esistono innocenti, ma solo colpevoli per i quali non si è dimostrata la colpevolezza. Aveva ragione. La tesi si è applicata anche

offendono. Voglio dire che noi rispettiamo la magistratura, ma la magistratura rispetti l'Italia. Queste sentenze sono riduttive e giustificazioniste: undici anni, per aver ucciso un maresciallo dei Carabinieri per strada, sono una vergogna.

ma anche coloro che li mandano a Fregene dalla nonna. Cerciello non può andare a Fregene dalla nonna. Sono lieto che almeno il maresciallo Manganaro, che mise un cerotto sugli occhi di uno di questi americani per impedire atti autolesionistici, sia stato recentemente assolto dalla magistratura, la quale stava forse condannando i carabinieri che arrestarono gli americani con più severità di quanta ne abbia usata per trattare gli americani. Amo l'America, ma depreco gli assassini che restano tali, anche se stanno dalla nonna a prendere il sole a Fregene. Vergogna per la magistratura italiana!

e, più in generale, alle criticità sofferte dall'istituto in questione, con particolare riguardo al sovraffollamento e alle carenze organiche e strutturali. Come evidenziato in sede di risposta ad interrogazioni di analogo tenore, al tema del sistema carcerario nazionale, così come al dramma dei suicidi di persone ristrette in carcere, questo Governo riserva la massima attenzione, con un costante impegno profuso dal Ministero della giustizia attraverso il Riguardo alla drammatica vicenda riportata, appare importante sottolineare alcune circostanze emerse dalla relazione del direttore dell'istituto penitenziario. Il detenuto era conosciuto dagli operatori e dal personale e, nel suo percorso, era riuscito a inserirsi gradualmente nella vita dell'istituto, partecipando alle attività comuni ed impegnandosi nell'attività lavorativa in qualità di addetto alla cucina, tanto che complessivo comportamento del ristretto non appariva poter degenerare in un tragico gesto. Accanto all'autonoma indagine dell'autorità giudiziaria, sono naturalmente in essere le doverose attività ispettive da parte del competente provveditorato regionale di Padova, proprio finalizzate alla esatta verifica di tutto quanto occorso nel periodo di detenzione sino al tragico evento; allo stato, come riferisce il DAP con nota dell'11 ottobre 2024, non sono ancora noti gli esiti dell'indagine ispettiva. Rispetto ai dati forniti dall'atto di sindacato ispettivo purtroppo si conferma che dal 1° gennaio al 9 ottobre 2024, presso gli istituti di pena del Triveneto si sono verificati sette eventi suicidari, di cui due presso la casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore. È altrettanto drammatico il dato nazionale rilevato dal 1° gennaio al 9 ottobre, periodo in cui si sono registrati 70 suicidi fra persone detenute. L'evidenza che emerge da questi dati ci impone il dovere di garantire l'incolumità personale dei soggetti affidati allo Stato nel periodo di esecuzione della pena, tutelandone anche la salute psicologica, in considerazione dello *shock* psicologico della privazione della libertà. Per tale ragione, uno dei fronti su cui il Ministero della giustizia è maggiormente impegnato è quello del potenziamento della rete di assistenza psicologica: esso è attuato sia con progetti di monitoraggio in corso da tempo, sia con un'integrazione concreta di ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro, relativamente al capitolo di spesa pertinente all'osservazione psicologica. Prosegue inoltre anche l'opera di reclutamento di adeguato personale specializzato, per rispondere alle crescenti esigenze riscontrate tra la popolazione carceraria. Per la prima volta è stata integralmente coperta la pianta organica dei funzionari giuridico pedagogici di circa 1.100 unità. Per psicologi e psichiatri il trasferimento dalla medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale richiede la collaborazione con gli organi sanitari regionali e territoriali, per l'erogazione dell'assistenza sanitaria presso gli istituti di pena. È in questo contesto che il Ministero sta costantemente interloquendo con la Conferenza Stato-Regioni, proprio per assicurare un tempestivo confronto sui temi dell'assistenza sanitaria, finalizzato all'attuazione di tutte le iniziative possibili a beneficio della popolazione carceraria. Anche sulla dotazione di risorse finanziarie il Ministero è intervenuto con determinazione. Per il 2024 le risorse a bilancio per i servizi di assistenza psicologica saranno circa 14 milioni di euro, quasi il triplo rispetto all'anno scorso. Si aggiunga che, atteso l'incremento dei fenomeni suicidari in ambito detentivo durante l'anno in corso, sono state individuate ulteriori strategie preventive: si sono sensibilizzate le articolazioni competenti a una revisione dei piani locali di prevenzione, prevedendo la convocazione dello *staff* multidisciplinare nell'immediatezza di un gesto autolesivo o di un tentativo di suicidio. Consapevoli del fatto che gli eventi critici si intrecciano con i problemi legati al cronico sovraffollamento carcerario, volgendo lo sguardo ai dati ultimi rilevati il 10 ottobre scorso,

In proposito deve ricordarsi che attraverso un costante monitoraggio dei dati relativi alle presenze detentive a livello nazionale, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento gestisce le procedure di riequilibrio, su scala nazionale, della popolazione detenuta: di recente, sono stati adottati provvedimenti deflattivi che hanno interessato proprio gli istituti del Triveneto con una maggiore presenza detentiva. Quanto all'assistenza sanitaria, si evidenzia che la casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore risulta essere dotata dei presidi fondamentali quali l'assistenza medica sull'intero arco giornaliero, e, nello specifico, specializzazione dermatologica, infettivologica, odontoiatrica, psichiatrica e presidio per tossicodipendenti. Oltre al monitoraggio delle presenze, grande attenzione viene posta alle criticità strutturali degli istituti penitenziari, tutti inseriti in un imponente e complesso piano nazionale di ristrutturazione e adeguamento, come già riferito in data 17 luglio 2024 in occasione di risposta al *question time*. Nello specifico, l'istituto penitenziario in esame, benché realizzato alla fine degli anni Venti del secolo scorso, è stato sottoposto a radicali lavori di ristrutturazione, con adeguamento di tutte le sezioni detentive alle prescrizioni di cui al DPR n. 230 del 2000. Allo stato, può affermarsi che non rilevano criticità degne di nota sotto il profilo edile, rimanendo l'attenzione focalizzata, invece, sul sovraffollamento detentivo; nell'ambito del piano nazionale degli interventi sulle infrastrutture carcerarie, è incluso il circondario del provveditorato regionale del Triveneto, con la previsione di nuovi posti detentivi in grado di attenuare l'attuale condizione di sofferenza anche della casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore. Sempre riferendomi ai dati riguardanti l'istituto veneziano, in relazione all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, risulta che, alla data del 9 ottobre 2024, il personale in servizio ammonta a 146 unità, con una carenza, dunque, di 32 unità rispetto alle previsioni organiche. Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (meno uno), e in quello dei sovrintendenti (meno 20), anche se, di contro, il ruolo degli agenti-assistenti risulta in esubero di quattro unità e l'area dei citati funzionari giuridico-pedagogici risulta avere cinque presenze effettive, su un organico di cinque unità. In tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto DAP, pone forte attenzione all'esigenza di garantire un efficace *turnover* del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati. Si rappresenta che, per integrare l'organico dei funzionari, il 18 dicembre 2023 è stato avviato il VII corso, relativo al concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo da distribuire a seconda delle vacanze. Si aggiunge che l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha previsto l'assunzione di ulteriori unità mediante scorrimento della graduatoria degli idonei concorsi per allievi commissari, che prenderanno servizio nel mese di maggio 2025. Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, si comunica che, si è concluso il corso per la nomina alla qualifica di vice ispettore, in esito al quale è stata assegnata alla casa circondariale di Venezia un'unità femminile. il 5 maggio 2024 ha preso avvio il corso di formazione per la qualifica iniziale di vice ispettore indetto per 411 posti, con presa di servizio effettiva a giugno 2025. Con riferimento al ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che l'amministrazione ha assegnato al reparto di Polizia penitenziaria della casa circondariale di Venezia tre unità maschili. Ulteriori 293 unità per la qualifica di vice sovrintendente saranno previste con il concorso interno bandito il 16 febbraio 2024. Ad ogni buon conto, si rappresenta che, per i ruoli di agenti e assistenti, l'8 luglio 2024, hanno assunto servizio negli istituti penitenziari 1.702 agenti, vincitori del concorso pubblico per 1.867 unità, indetto il 31 marzo 2022. Inoltre, il 22 luglio 2024 è iniziato il corso di formazione per per 1.713 agenti vincitori di concorso, che assumeranno servizio nei vari istituti penitenziari nel mese di febbraio 2025. Infine, con provvedimento del direttore generale del 6 marzo 2024, è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 2.568 allievi agenti, attualmente in corso.

è persino peggiorata, Infatti, dopo il suicidio del detenuto di San Donà di Piave presso il carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia ad inizio ottobre vi è stato un altro, ennesimo, suicidio, questa volta a Vicenza, evidenziando quanto il sistema ormai sia al collasso. Come lei ha ricordato e come riporta l'ultimo *report* del Garante dei detenuti, sono già 72 le persone che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno: un dato in crescita rispetto al 2023. Per quanto riguarda la casa circondariale di Venezia, essa versa davvero in condizioni drammatiche, nonostante gli sforzi di iniziativa encomiabile della direzione, degli operatori e degli agenti. A Santa Maria Maggiore ci sono 257 (fino a ieri, lei oggi ha detto 258) detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 159 persone: 100 detenuti in più oltre la capienza prevista, con un tasso di sovraffollamento che continua a crescere e che oggi ha superato il 61 per cento. È il secondo dato più alto in Veneto, secondo solo alla casa circondariale di Treviso e fra i primi in Italia, che in questi giorni ha toccato il massimo storico. cento di detenuti di origine straniera, manca il mediatore culturale di lingua araba, così come manca un luogo dedicato ai culti diversi da quello cattolico. I corsi di alfabetizzazione riguardano una minoranza della popolazione detenuta che non parla italiano. Le attività lavorative riguardano solo 70 detenuti, di questi solo il 10 per cento impiegati in attività lavorative gestite da terzi. Non sono garantiti tre metri quadrati calpestabili, non è garantita la divisione fra adulti e giovani adulti. «Antigone» e «Nessuno tocchi Caino» segnalano inoltre lo scarso livello di manutenzione infrastrutturale e l'assenza di spazi per le socialità adeguatamente arredati. Nel 2024, l'ha ricordato anche lei, ci sono stati oltre 100 casi di autolesionismo, 12 tentati suicidi, 2 suicidi; i sindacati di Polizia segnalano 60 eventi critici nell'ultimo anno, decine di aggressioni ai danni del personale, tre in in occasione di un'ultima rivolta nel luglio di quest'anno. La Polizia è al 70 per cento del personale previsto e quindi sotto organico: una situazione che non è affatto migliorata, anzi è peggiorata a seguito del decreto carceri, anche perché l'immissione in ruolo del personale è prevista su più anni e con un effetto che possiamo dire verrà neutralizzato dalle uscite per pensionamento e dimissioni. E non è l'unica lo abbiamo detto in tante occasioni - lacuna di un decreto che non ha dato risposte all'emergenza carceri presente nel nostro Paese. Anche per quanto riguarda le carenze dell'area educativa e sanitaria, la situazione è davvero molto complicata. Sono presenti solo cinque educatori, uno ogni 50 detenuti. Sono garantite solo cinque ore di presenza dello psichiatra a settimana, tre per lo psicologo: questo su una platea che, nel corso dell'ultima visita, «Nessuno tocchi Caino» ha detto essere una platea in cui il 98 per cento dei detenuti fa uso di psicofarmaci e stabilizzanti dell'umore. È un quadro davvero drammatico e non c'è nessuna enfasi particolare in tutto quello che ho detto. Purtroppo, l'approccio securitario, muscolare e sanzionatorio, sulla spinta di un panpenalismo che ha inventato nuovi reati e ha inasprito le pene, rischia, invece di alleggerire il sovraffollamento, di far esplodere le carceri. Questo è quello che sta succedendo. Se si pensa che il carcere sia l'unica risposta che si può dare, veramente non si è capito nulla della società italiana. Occorre investire sul reinserimento sociale, sul fine rieducativo della pena, sul lavoro, sulla formazione, sugli organici: tutto questo non è tempo perso. Bisognerebbe prendere la strada delle misure alternative in un quadro di sicurezza sociale complessiva, perché dovremmo occuparci e preoccuparci anche del momento successivo all'uscita dal carcere, per evitare la recidiva e che la condanna ad una vita illegale permanente non abbia possibilità di riscatto. Al carcere di Santa Maria Maggiore faremo una nuova visita nei prossimi giorni e chiederemo interventi per migliorare la qualità della vita della popolazione carceraria e degli operatori. Continueremo costantemente a monitorare la situazione del sistema penitenziario in Veneto e a Venezia, perché facciamo nostro il pensiero di chi ha detto che il grado di civiltà di un Paese si misura anche dalle condizioni delle sue carceri.

finestra") sui criteri per l'erogazione del *bonus* aggiuntivo alle tredicesime, Il *bonus* è erogato sia alle famiglie di conviventi, sia alle famiglie monogenitoriali; alle prime, è erogato se sono sposate, hanno un figlio, un coniuge a carico e un reddito che non supera i 28.000 euro lordi. Ai coniugati sono equiparate le coppie di conviventi soltanto se registrate come unioni civili. I nuclei monoparentali sussistono qualora il figlio sia stato affidato a un solo genitore oppure quando un genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio. In sostanza, il *bonus* va alle famiglie tradizionali di sposati, dove un coniuge (nella maggior parte dei casi la donna) non ha un'occupazione. Questo è in netto contrasto con le dichiarazioni del Governo e i *bonus* finalizzati a incentivare l'occupazione femminile. Va alle famiglie monoparentali se hanno l'affidamento esclusivo, che taglia fuori la maggior parte dei genitori separati giudizialmente, oppure nei casi in cui l'altro genitore è venuto a mancare o è rimasto sconosciuto. Tutto ciò nonostante le note difficoltà delle famiglie monogenitoriali, all'interno delle quali un solo reddito, spesso senza il contributo dell'altro genitore, non è sufficiente a coprire le spese della vita quotidiana. Peraltro, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, in Italia (con l'unica eccezione del Sud Tirolo) non esiste neanche l'istituto dell'anticipazione del contributo al mantenimento da parte dello Stato. L'impressione è che i criteri per l'accesso al *bonus* siano formulati per restringere il più possibile la platea dei destinatari, disincentivando le donne a ricercare un'occupazione e gli uomini a riconoscere i propri figli. Tutto ciò premesso, si chiede al Ministro in indirizzo: se voglia indicare il numero effettivo dei destinatari del contributo statale illustrato in premessa, che non può essere quello di 1,1 milioni di lavoratori indicato nella relazione tecnica relativa alla misura, in quanto tiene conto solo del dato reddituale; se voglia spiegare quale sia il ragionamento che sta alla base della determinazione dei criteri per l'accesso alla misura; se ritiene che tali criteri siano da considerarsi valevoli anche per le future elargizioni di contributi statali a lavoratori e famiglie.

ha previsto per l'anno 2024 il riconoscimento di un'indennità *una tantum*, nella misura massima di 100 euro (il cosiddetto *bonus* Natale), da corrispondere insieme alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti. Considerati i requisiti necessari per la sua erogazione, gli interroganti lamentano che il *bonus* in argomento venga di fatto riconosciuto solo alle famiglie tradizionali monoreddito e solo ad alcune categorie di famiglie monogenitoriali, di fatto contravvenendo gli intendimenti del Governo volti, ad esempio, a incentivare l'occupazione femminile. Tanto premesso, gli interroganti chiedono chiarimenti sul numero effettivo dei percettori, quali siano stati i criteri di scelta dei parametri individuati per l'accesso al beneficio e se tali criteri saranno ritenuti valevoli anche per eventuali successive elargizioni. Osservo che l'indennità introdotta dalla disposizione è destinata, in particolare, ai lavoratori a più basso reddito. Per questo motivo, si inserisce nel solco di un impianto normativo già esistente e collaudato; prevede un trattamento integrativo che spetta a determinate condizioni capienza dell'imposta lorda e limite di reddito a 28.000 euro - offrendo un sostegno per il coniuge a carico riconosciuto tramite una specifica detrazione e una particolare attenzione verso specifici nuclei monogenitoriali (ai quali è consentito fruire in dichiarazione, per il figlio, della più favorevole detrazione per il coniuge). Si è scelto di operare in base a tali criteri al fine di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari, compatibilmente con le disponibilità di bilancio per l'anno 2024. Alla luce di quanto esposto, si conferma la stima di 1,1 milioni di beneficiari, effettuata in base alle dichiarazioni dei redditi sulle quali è stata verificata la presenza di tutti i requisiti: limite di reddito, presenza dei carichi familiari necessari (figlio a carico o più coniugi a carico, oppure figlio come coniuge), capienza dell'imposta lorda ai fini del trattamento integrativo. In particolare, si specifica che il numero dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a 28.000 euro è di circa 16,5 milioni, di cui quelli con imposta lorda capiente, ai fini del trattamento integrativo, sono circa 12,3 milioni. In ultimo, si fa presente che i criteri individuati dalla disposizione, nel solco di quanto originariamente previsto dallo schema di decreto delegato recante revisione del regime impositivo dei redditi, sono stati calibrati esclusivamente per la misura in argomento, non risultando vincolanti in relazione a eventuali future iniziative in favore di famiglie e lavoratori.

perché si istituisce un *bonus* che ricevono solo donne che non hanno occupazione o solo famiglie monogenitoriali in cui il padre non ha riconosciuto il figlio. Mi sembrano criteri veramente assurdi che non hanno alcun senso, che restringono

la manovra di quest'anno sarebbe stata molto dura e con sacrifici per tutti, e dopo la sollevata di scudi della sua maggioranza, compreso il suo partito, pensavo che, per doverla rivedere, avrei dovuto chiamare «Chi l'ha visto?». Mi fa invece piacere vederla in

leggiamo che c'è un riallineamento delle aliquote *diesel* e benzina e, quindi, si è ipotizzato che ci potesse essere un aumento delle accise. Lei stesso ha parlato dell'introduzione dell'IMU per le case che avevano ottenuto il superbonus. Insomma, si sono fatte varie ipotesi. Lei ieri ha fatto una bellissima conferenza stampa dove, nell'elencare gli elementi per cui in teoria dovrebbero arrivare delle nuove entrate, ha parlato della famosa tassa sulle banche.

è venuto da molto in basso avendo dovuto studiare molto per arrivare alla posizione in cui si trova è molto attento a leggere le carte. Lei sa benissimo che quello è un anticipo di spesa,

Sono soldi insufficienti per la spesa sanitaria. Voi siete bravissimi a comunicare: avete subito detto che le banche finanzieranno la sanità, ma parliamo di 2,7 miliardi e la sanità costa 332,6 miliardi.

Prima di tutto, con riferimento alla annosa questione sollevata rispetto all'annunciato riallineamento delle aliquote delle accise per *diesel* e benzina, ultima analisi rispondono a un preciso obbligo rispetto all'impostazione assunta in sede europea

per il preciso obbligo e impegno del PNRR - il Governo rimetterà al Parlamento poi la scelta definitiva, come è giusto che sia - abbiamo detto che è corretto l'allineamento, che potrà essere graduale potrà significare, quindi, l'aumento dell'accisa sul gasolio. Ma evidentemente la diminuzione dell'accisa sulla benzina nelle forme stabilite, appunto, dal Parlamento risponde a una precisa politica che - come a tutti è noto si sta anche rivedendo in sede europea, e su cui chi parla, e comunque questa maggioranza, non è mai stato d'accordo. Si è fatta anche molta polemica rispetto all'aumento delle tasse sulla casa. È assolutamente falso. Ma credo che chiunque abbia un minimo di esperienza sappia perfettamente che chiunque fa un'operazione di ristrutturazione edilizia, tanto più quella addirittura pagata dallo Stato, ha un preciso obbligo: aggiornare i dati catastali. Naturalmente, noi siamo tenuti - e lo faremo - a verificare l'aggiornamento dei dati catastali e quelli di coloro che le case non le hanno mai dichiarate. Per quanto riguarda la possibilità di finanziare la sanità e tutte le misure che abbiamo annunciato, è il frutto del nostro lavoro, dei dati del 2024, che sono giudicati positivamente, magari non in quest'Aula dall'opposizione, ma da tutti gli osservatori economici nazionali e internazionali, e i dati oggettivi - anche oggi quelli dello *spread* - ci confortano. Abbiamo creato le condizioni di finanza pubblica per poter abbassare le tasse ai redditi medio-bassi. Avevamo detto che lo avremmo fatto, continuiamo a farlo e lo abbiamo reso strutturale.

come Italia Viva, che le tasse vengono diminuite. In realtà, sa chi pagherà la manovra? Non la pagheranno né le banche, né le assicurazioni, né i potenti che ci sono in questo Stato, ma la pagheranno semplicemente i cittadini che già pagano le tasse. Voi avete deciso di fare una diminuzione delle detrazioni favorendo una vostra scelta - le famiglie numerose, che sono il 3,7 per cento della popolazione italiana, facendola pagare ai *single*, ai nonni, alle famiglie con figli adulti, che si vedranno semplicemente tagliati

il ceto medio (cioè insegnanti, infermieri e impiegati) abbia il diritto di essere rispettato: non solo in campagna elettorale, ma anche nella vita reale.

non sono fessi e capiscono che, in sostanza, ancora una volta a pagare sono solo e sempre gli stessi, perché chi in questi anni ha guadagnato molti soldi non tirerà fuori un euro. A mio

Quest'anno abbiamo anche chiesto un contributo significativo a banche e assicurazioni. Devo dire con ironia che l'anno scorso ci contestavate il fatto che abbiamo fatto una tassa sugli extraprofitti e non hanno versato un euro, quest'anno ci dite che versano gli euro, ma non abbiamo fatto la tassa. Il risultato è che noi abbiamo la disponibilità, grazie alla quale possiamo incrementare il Fondo sanitario nazionale a favore degli interventi nella sanità

Tutte le contestazioni che abbiamo avuto in merito all'aggiornamento dei dati catastali sono dovute al fatto che vogliamo andare a recuperare l'evasione e non aumentare le rendite catastali a tutti i cittadini che giustamente hanno una casa e hanno fatto il loro dovere. Ritengo che il comportamento del nostro Governo non sia in questo senso meritevole di biasimo. Continueremo in questa direzione e credo che i dati ci diano ragione. intervenire in replica il senatore De Cristofaro,

a reti unificate, se posso dire così, a tutti i giornali, che bisogna questa volta mettere in campo una tassa per i profitti in eccedenza, in particolare di quelli delle banche. Ha altresì richiamato l'articolo 53 della Costituzione,

decine di milioni di italiani si sono molto impoverite e in pochissimi si sono molto arricchiti attraverso gli extraprofitti. Lei ci aveva fatto comprendere che, finalmente, in questo modo quest'anno si sarebbe messo mano a tale elemento di diseguaglianza.

di destra sociale, ha fatto sì che la presunta e giusta tassa sugli extraprofitti diventasse invece semplicemente un anticipo di cassa che verrà recuperato. Non è vero che con questo anticipo di cassa si

uno stanziamento iniziale di 1.575 milioni. In questa legislatura siamo riusciti a ottenere un risultato davvero importante e insperato alla vigilia, tanto che l'indennizzo che è stato corrisposto ai truffati delle banche è salito dal 30 al 40 per cento del costo delle azioni che erano state acquistate. Credo sia un successo che voglio condividere con lei, di cui i risparmiatori che stanno ascoltando devono essere consapevoli. La commissione tecnica ha concluso i lavori il 31 ottobre dell'anno scorso. Da tutti i dati in nostro possesso è risultato un residuo di cassa. La prima domanda che io le formulo è proprio volta a conoscere l'ammontare di questo residuo di cassa. chiacchiere - diciamo così - le stime di chi si è occupato di questo argomento lo indicano in circa 250.000 euro. Ciò detto, io non vengo oggi a chiederle la distribuzione di questo residuo di cassa perché immagino,

Governo che si era impegnato a valutare - l'opportunità di istituire la possibilità per i risparmiatori, che hanno commesso errori formali o procedurali, di veder riesaminata la loro posizione. Le spiego anche, signor Ministro, da che cosa nasce questo mio impegno, particolarmente assiduo su questo tema. Il mio ex professore di educazione fisica del liceo ha commesso un errore: di fronte al portale, nel momento in cui ha inserito i dati - e qui ho le parole testuali che arrivano dalla Consap - ha presentato domanda di indennizzo, indicando di essere titolare di 439 azioni;

l'impossibilità di modificare questa domanda introduttiva, fa sì che sia rimasto pretermesso. Lui, così come altri, ha commesso degli errori; credo però che di fronte a queste situazioni sia possibile - e io ho formulato l'ipotesi che il Governo valuti tale possibilità - aprire un termine per adire l'arbitro delle controversie finanziarie, che è una procedura *light*, poco costosa, per cui non occorre neppure l'avvocato. Ciò consentirebbe a certe posizioni (ripeto: errori formali

Signor Presidente, senatore Zanettin, richiamo la vicenda a beneficio di tutta l'Assemblea, perché lei la conosce meglio di tutti. Il termine per la presentazione delle istanze per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prorogato più volte, è scaduto il 18 giugno 2020. È stato consentito ai risparmiatori che avevano presentato istanze incomplete di regolarizzarle entro il 1° maggio 2022; la Commissione tecnica incaricata dell'esame delle richieste, dopo numerose proroghe, ha concluso i lavori il 31 ottobre del 2023. Nel corso degli anni 2022 e 2023, la Commissione tecnica del FIR ha istruito 144.871 pratiche, riesaminando tra l'altro in sede di autotutela 1.633 istanze di revisione. Sono state accolte 134.136 istanze, erogando complessivamente l'importo di 1.353.832.529 di 1.353.832.529 a 129.899 risparmiatori. Per quanto riguarda le controversie giudiziarie promosse, relativamente a richieste di indennizzo non accolte, sono state conservate in bilancio le somme necessarie per dare copertura alle eventuali erogazioni conseguenti all'esito delle stesse. Ciò posto, in conseguenza del completamento dell'attività del fondo entro il detto termine del 31 ottobre 2023, la dotazione di bilancio residuo del FIR è divenuta economia di bilancio dello Stato e, pertanto, al di là degli accantonamenti per le cause pendenti, non sussistono allo stato ulteriori risorse. all'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno citato - attesa la specificità e l'eccezionalità della disciplina del FIR, che al momento della sua definizione fu oggetto di approfondita interlocuzione con gli uffici della Commissione europea al fine di evitare contestazioni in tema di aiuti di Stato sono in corso approfondimenti sull'opportunità di intervenire per risolvere definitivamente il contenzioso ancora in corso. Per quanto concerne le domande respinte per ragioni procedurali, come ho appena illustrato, è stata già consentita la possibilità di regolarizzarle dopo la scadenza del termine del 2020, mentre ulteriori fattispecie di remissione in termini per irregolarità meramente formali richiederebbero l'adozione di ulteriori specifici interventi normativi, dotati, per le ragioni che ho illustrato, di autonoma copertura finanziaria, che ovviamente dovranno essere valutate nel quadro attuale di finanza. Signor Presidente, sono solo parzialmente soddisfatto della risposta, nel senso che il fatto che ci siano state delle proroghe non risolve il problema, perché questi risparmiatori si sono accorti dell'errore solo quando gli è stata data la risposta e il termine era già scaduto per fare ricorso. Dal punto di vista Dal punto di vista tecnico la sua risposta appare carente, perché queste persone hanno appreso solo in una fase successiva che avevano commesso degli errori. Poi, resto abbastanza sorpreso del fatto che, al di là del disaccantonamento per i contenziosi in essere,

i risparmiatori e la tutela dei truffati dalle banche. Prendo atto della disponibilità del Ministro a ragionare su questo tema. Io ho presentato diversi emendamenti, come lei ben sa, ai vari disegni di legge e veicoli normativi che sono transitati qui in Parlamento e fino ad oggi, effettivamente, sono stati tutti dichiarati inammissibili, improcedibili e quant'altro. Spero che nel dialogo costante che abbiamo avuto con lei e con la dottoressa Perrotta in questi anni si possa trovare la strada e la scappatoia per risolvere questi che sono casi concreti di vita reale, dietro i quali si celano

Signor Presidente, signor Ministro, sottopongo alla sua attenzione una situazione emergenziale che si sta verificando nel territorio del Trentino in relazione alla convivenza con l'orso bruno. Il progetto Life Ursus che fu promosso nel 1999 dal parco naturale Adamello Brenta, insieme alla Provincia autonoma di Trento e ad ISPRA, si è concluso con successo nel 2004, anche grazie ad accordi operativi con le quattro province confinanti e con l'Associazione dei cacciatori trentini. Purtroppo, se la risposta degli orsi ha realizzato gli auspici dell'incremento numerico del nucleo di orsi già presenti, altrettanto non si può dire di quella dell'uomo. Non risultano infatti essere state implementate nel corso di questi decenni le misure previste dal progetto originario: a) la dotazione di bidoni della spazzatura anti orso per evitare che, attratti da cibo facile, si avvicinino all'abitato; b) la piantumazione di alberi da frutto nelle zone più interne per indurne la stabilizzazione lontano dall'abitato; c) la creazione di corridoi faunistici per consentire l'esplorazione del territorio e l'espansione per il ricongiungimento di tutte le popolazioni alpine; d) la campagna informativa ed educativa dei residenti, dei turisti e degli avventori; la pluridecennale inerzia amministrativa ha fatto sì che gli orsi si avvicinassero ai centri abitati, attratti dall'odore dei resti di cibo nella spazzatura e che così divenissero confidenti con l'uomo, creando i presupposti per il verificarsi di situazioni di pericolo più che occasione di danneggiamenti. La cronaca e i mass media riportano gli episodi in cui alcuni orsi sono stati coinvolti in situazioni di confidenza e di contatto, anche violento, con esseri umani, dalle dinamiche tuttora da accertare nel dettaglio; nel tempo sono stati trovati morti, catturati, uccisi o allontanati in strutture diversi orsi; in data 12 ottobre 2024 l'interrogante si è recata in visita preannunciata al centro di recupero della fauna alpina di Casteller, dove attualmente sono rinchiusi i due orsi e ha verificato personalmente che il luogo non appare idoneo a garantire condizioni di vita compatibili con la loro natura di animali selvatici: sono costretti in spazi troppo ristretti (0,3 ettari), privati degli stimoli naturali, confinati in condizioni punitive e penalizzanti per un periodo di tempo troppo lungo e ben lungi dall'avere una valenza riabilitativa; risultano depositati numerosi progetti di autorevoli associazioni ambientaliste per favorire e promuovere il rispetto e la convivenza con la fauna selvatica da colloqui con la cittadinanza e con le associazioni del territorio emerge che è attualmente in corso una strage silenziosa, messa in atto con sistemi di bracconaggio strisciante e abbandono di esche avvelenate, che peraltro mietono vittime tra tutta la fauna indistintamente, se il Ministro in indirizzo, al fine di tutelare l'orso bruno quale bene indisponibile dello Stato, intenda avviare iniziative, di concerto con i competenti enti, per la tutela e la salvaguardia della popolazione degli orsi bruni presente nella provincia di Trento, con particolare riferimento alla creazione di corridoi faunistici per la distribuzione degli orsi nei territori limitrofi, per il ricongiungimento con altre popolazioni, piantumazione di alberi da frutto, fornitura di bidoni anti-orso immediata e interventi di educazione. Domando se intenda prevedere appositi fondi per finanziare ulteriori specifici progetti, anche sperimentali, di concerto con concerto con i competenti enti territoriali, che possano conciliare la conservazione della specie e garantire la sicurezza pubblica, compreso l'ampliamento delle aree destinate al contenimento riabilitativo della fauna selvatica presso il Casteller ciò dovrebbe avvenire realizzando aree di contenimento degli orsi confidenti allo scopo di rieducarli alla selvaticità per poi reinserirli in natura, evitando il trasferimento degli orsi in parchi zoo, all'estero o in Italia, che provocherebbero immani sofferenze psichiche e fisiche. Chiedo inoltre se il Ministro intenda attivare uno specifico tavolo tecnico per la trattazione delle problematiche riguardanti la popolazione plantigrada, coinvolgendo Regioni e Province autonome, enti competenti, associazioni ambientaliste e rappresentative delle categorie, al fine di garantire il rispetto degli spazi destinati alla fauna selvatica, attivandosi affinché siano disincentivati comportamenti umani che possono interferire con la vita selvatica degli orsi e mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha promosso e condiviso, con tutte le Regioni e le Province autonome interessate, il Piano d'azione per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali, il cosiddetto Pacobace, che guida le azioni di conservazione della specie nel rispetto del vigente quadro normativo nazionale e unionale. Lo scorso anno, nel contesto dei confronti tecnici sul tema promossi dal MASE, l'ISPRA ha prodotto uno specifico rapporto con l'obiettivo di definire strategie di intervento e per la prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica legati alla presenza degli orsi. Nel rapporto, l'ISPRA riferisce che spesso le condotte potenzialmente pericolose sono la conseguenza di comportamenti umani non adeguati alla presenza della specie nel territorio, per cui è prioritario agire su tali fattori, oltre che sugli individui potenzialmente pericolosi. In ogni caso, le strategie di intervento devono tener conto di tutte le misure possibili, dai corridoi faunistici alla fornitura di bidoni anti-orso. Al tempo stesso, sono in corso presso ISPRA valutazioni tecniche sull'attuabilità dei programmi di sterilizzazione degli esemplari, da considerare come metodologia alternativa al mero abbattimento selettivo, che devono valutare attentamente le ricadute in chiave demografica sulla specie, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. È alquanto inesatto, quindi, parlare di inerzia amministrativa dinanzi a tali azioni nazionali e alle attività regionali. Basti pensare a tutte le attività e ai finanziamenti messi in campo dalla Provincia autonoma di Trento dall'avvio del progetto Life Ursus, dai progetti di comunicazione alle attività di messa in sicurezza dei rifiuti organici con dispositivi anti-orso, alla costituzione di tavoli che vedono la partecipazione attiva di associazioni ambientaliste ed esperte in tale ambito. Un'ultima specifica faccio sulla struttura di di Casteller, citata dagli interroganti. Va rimarcato che essa mantiene la sua funzione di struttura di primo ricovero, temporalmente limitato. Anche sulla base di specifiche analisi condotte negli anni passati, la realizzazione delle aree di contenimento degli orsi confidenti non risulta percorribile, poiché non è possibile rieducarli alla selvaticità

Signor Ministro, non sono soddisfatta della sua risposta, in quanto non mi sembra che in questo modo venga tutelato il sentimento

tanto vale che vengano uccisi, come dicono in tanti, anche delle associazioni ambientaliste, piuttosto che fargli sopportare certe condizioni. Vorrei focalizzarmi però su un particolare: la creazione dei corridoi faunistici non viene per il momento implementata.

del resto del Governo affinché vengano stanziati i fondi per la creazione dei corridoi faunistici, che non dobbiamo immaginarci come dei ponti sopraelevati, tipo Stretto di Messina (dove ci sono 14 miliardi stanziati). Qui stiamo parlando semplicemente di pulire i cunicoli sotterranei attualmente esistenti. È un investimento di bassa caratura, che però risolverebbe un problema, perché, consentendo a quegli animali di spostarsi e di accedere a un territorio più vasto,

senatrici e senatori, signor Ministro, il suo compito dovrebbe essere anzitutto quello di difendere la sua funzione di Ministro dell'ambiente in un Governo contro la sostenibilità, che barcolla tra il negazionismo del caos climatico e il fare spallucce, rinviando o aggirando gli impegni. Lo ha detto qui due giorni fa la presidente Giorgia Meloni. Eppure, aumentano le patologie in un pianeta sempre più ostile per la specie umana e, invece, più comodo per zanzare e topi; aumentano gli eventi climatici estremi e agli alluvionati voi dite di farsi un'assicurazione, e cioè, di arrangiarsi, perché non stanziate risorse sufficienti. Lo stesso vale per l'agricoltura, colpita da siccità e da malattie generate proprio dagli squilibri climatici. I ristori, se va bene, sono pari al 4 per cento e migliaia di imprese chiudono. Insomma, non volete curare, non volete prevenire e vi affidate alla Divina Provvidenza o al "si salvi chi può". Questa interrogazione, signor Ministro, lo dimostra. Vantate di essere in linea con lo stato di avanzamento del PNRR, ma omettete di dire che avete speso un quarto dei fondi disponibili (53 miliardi su quasi 200) e che più di un quarto di questi è proprio il *superbonus* in edilizia. Esso è per voi il male assoluto quando dovete giustificare i soldi che non ci sono per sanità e lavoro, ma diventa il bene assoluto quando vi serve a dire che siete in linea con il PNRR e che i dati sull'occupazione sono in crescita - e ci mancherebbe pure, con risorse che sono 10 volte il piano Marshall e che voi nemmeno volevate - omettendo di aggiungere che è proprio grazie all'edilizia che aumenta il lavoro povero. La verità è che siete molto indietro, in particolare nel PNRR destinato proprio alla transizione ecologica e alle 6 misure relative, rispettivamente, allo sviluppo del biometano, al rafforzamento della *smart grid,* al potenziamento del parco autobus regionale, all'industria delle batterie, alla capacità delle rinnovabili, agli investimenti in infrastrutture idriche primarie e per le quali corrispondono circa 3,1 miliardi. Le spese effettivamente ammontano a 250 milioni, pari solamente, quindi, all'8 per cento delle risorse previste.

In relazione ai quesiti posti si rappresenta in via preliminare che, in base alle informazioni fornite dalla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla data attuale, ha rendicontato tutti gli obiettivi di propria competenza, nel pieno rispetto del cronoprogramma procedurale del PNRR, e ha assicurato un confronto costante con la Struttura di missione PNRR e la Commissione europea, assicurando al contempo l'aggiornamento del sistema ReGiS, dal quale non emergono criticità in ordine al raggiungimento di tutti gli obiettivi connessi alle singole misure di competenza. È altresì opportuno rappresentare che la metodologia del calcolo indicata dall'interrogante non risulta coerente con quella adottata. Difatti, il quadro complessivo dell'avanzamento della spesa deve essere necessariamente letto attraverso la tipicità di un programma basato sulla *performance*, per il quale non è corretto effettuare raffronti lineari circa le spese sostenute, come se tutti gli investimenti dovessero avere la medesima modalità e tempistiche di attuazione. È dunque inesatto considerare come base di calcolo per la determinazione della percentuale di avanzamento finanziario misure le cui *milestone*, consistenti nell'aggiudicazione dei progetti, sono ancora da conseguire nel rispetto della *deadline* prevista dal piano. A dimostrazione che il processo di liquidazione è entrato a pieno regime, si segnala che il numero di operazioni di trasferimento di risorse - effettuato nei primi nove mesi del 2024 - è stato oltre sei volte superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con riferimento ai profili attinenti all'avanzamento finanziario del Piano, le misure di competenza del MASE attivate, rispetto alla relativa dotazione assegnata, mostrano già uno stato di avanzamento ben superiore a quello evidenziato dall'interrogante, attestandosi al 59,38 Per i dettagli sui singoli investimenti, collega, le lascio eventualmente la tabella che riguarda *smart grid*, biometano, impianti di gestione dei rifiuti, infrastrutture di ricarica: ciò proprio per la massima trasparenza.

relative alle misure di competenza, e una specifica pagina è dedicata all'aggiornamento su base semestrale dello stato d'avanzamento di tutti gli investimenti del PNRR di competenza. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Fina, *(PD-IDP)*. Gentile Ministro, ma se non sono soddisfatti milioni di italiani e di italiane, possiamo essere soddisfatti noi? Qui parliamo non di astruse valutazioni di finanza pubblica, metodi di calcolo o di vuote schermaglie ideologiche, ma di questioni concrete, della vita quotidiana di famiglie e imprese, di bollette, in un Paese nel quale il costo dell'energia è il più alto d'Europa (ad agosto abbiamo pagato 128 euro a megawattora contro i 91 della Spagna, gli 82 della Germania, i 54 della Francia). Parliamo di povertà, e non solo della povertà di coloro che per colpa vostra non possono più accedere a misure di sostentamento minimo, non solo di chi lavora ed è povero, non solo di chi rinuncia alle cure, ma anche dei poveri energetici, di chi non ha soldi per scaldarsi in inverno e di chi non ha soldi per condizionare l'aria rovente in estate. Parliamo di marginalità, di chi vive in montagna, di chi vive in abitazioni energeticamente inefficienti. Parliamo di lavoro, di crisi dell'*automotive*, che è il principale settore industriale di questo Paese e che rischia di perdere migliaia di posti di lavoro. Parliamo del Paese reale, in particolare di quella parte del Paese che fa più fatica o che fa impresa, ma che non riesce a essere competitiva e chiude. Parliamo dell'Italia intera, insomma, danneggiata irreparabilmente dai vostri ritardi.

finestra") *(FdI)*. Signor Ministro, in un mondo sempre più colpito dai cambiamenti climatici, è imperativo adottare soluzioni concrete per evitare sprechi, ridurre il consumo e proteggere le fonti e le infrastrutture idriche al fine di garantire il futuro sostenibile per le generazioni future. Il Governo Meloni ha già mosso passi significativi attraverso il decreto siccità: un provvedimento volto a promuovere la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire un approvigionamento idrico sicuro. Lo scorso aprile i Ministri del G7 su clima, energia e ambiente, guidato dalla Presidenza italiana, hanno assunto per la prima volta un impegno specifico riguardo alla gestione delle risorse idriche, riconoscendo l'importanza vitale dell'acqua non solo come risorsa naturale, ma anche come diritto fondamentale per ogni essere umano. In particolare, è stata istituita una coalizione del G7 per l'acqua, con il compito di affrontare la crisi idrica globale e portare il tema all'attenzione dell'agenda politica internazionale. Pertanto, le chiediamo con questa interrogazione quali ulteriori iniziative intenda porre in essere al fine di promuovere politiche efficienti in materia di questione idrica, in vista della COP29 sui cambiamenti climatici, che si svolgerà in autunno in Azerbaijan, in particolare a Baku.

Al fine di identificare obiettivi e strategie comuni, è stata promossa una coalizione del G7 per l'acqua, concepita secondo un modello di *governance* che consenta all'Italia di giocare un ruolo di regista nella promozione delle azioni internazionali sul tema, incluse quelle relative alla sensibilizzazione e all'educazione per l'uso razionale delle risorse idriche. Pertanto, il 30 settembre scorso ho inviato un messaggio ai Presidenti e segretari esecutivi delle tre COP (COP clima, COP biodiversità e COP desertificazione) richiedendo di porre una maggiore attenzione alla risorsa idrica all'interno dei loro programmi di lavoro: tutto ciò al fine di addivenire, anche mediante la cooperazione transfrontaliera, a soluzioni efficaci e inclusive per rafforzare le politiche idriche e promuovere la resilienza alle sfide globali, a partire dalla gestione integrata delle risorse. L'intento è stimolare un confronto sulla gestione idrica a tutti i livelli, perché sia sostenibile, inclusiva ed adattiva, per bacini acquiferi sotterranei, in linea con la Conferenza di New York del 2023 e la recente strategia su acqua e servizi igienico-sanitari, adottata in occasione dell'ultimo Forum politico di alto livello. Ricordo, inoltre, che, tra il 2 e il 13 dicembre prossimo, si terrà a Riyad la 16a sessione della Conferenza delle Parti nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione: essa rappresenterà un foro privilegiato nell'ambito della quale discutere sulle sfide contingenti contro la desertificazione e per la salvaguardia delle risorse idriche. Segnalo, infine, che il Ministero, proprio in considerazione dell'importanza riservata al tema delle risorse idriche, intende farsi promotore del primo Forum euromediterraneo sull'acqua.

ragazza curda iraniana di ventisette anni: fuggita dall'Iran per le minacce che stava subendo, oltre che per il fatto di essere di una minoranza che in Iran è particolarmente perseguitata, arrivata a Crotone il 31 dicembre dell'anno scorso. Non le ha portato fortuna essere arrivata l'ultimo giorno dell'anno, perché all'inizio di quello successivo si trovava in carcere, accusata di essere la scafista.

nel nostro Paese. Tuttavia, nonostante l'assenza di evidenze, di testimonianze, di possibili ragioni per cui lei debba continuare a rimanere in carcere - è al secondo sciopero della fame e le sue condizioni di salute non sono certo ottimali - noi continuiamo a sapere che è lì. Non è l'unica: un'altra ragazza iraniana è, attualmente, agli arresti domiciliari sempre in Calabria, anche lei accusata di essere scafista, quando invece era l'autrice di una denuncia nei confronti di altre persone presenti sulla barca, che sono quelli che, di fronte all'essere stati denunciati di molestie, l'accusano invece di essere la scafista. Maysoon Majidi ha scritto al Presidente della Repubblica delle parole che vorrei riproporvi: venuta in Europa con la speranza di trovare una nuova casa e una nuova vita in una Nazione in cui diritti umani, libertà e dignità dell'individuo hanno valore. Prega di non essere lasciata sola, la nostra azione può fare la differenza tra speranza e disperazione, tra libertà e prigionia. E si rivolge al Presidente della Repubblica e al popolo italiano con la speranza che la sua voce venga ascoltata e che la sua situazione venga risolta con giustizia e umanità. Ho svolto questo intervento perché io penso che lei non vada lasciata sola e che, anche di fronte alle tante traversie che oggi segnano la geopolitica, non ci si può dimenticare di quelle ragazze e ragazzi iraniani che continuano a lottare per un futuro futuro migliore. Non possiamo dimenticarci di persone che stanno lottando per un mondo libero: quello nel quale noi viviamo, ma che forse vorremmo anche per gli altri. Per questo penso che